***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno***

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Prima di dare inizio ai lavori, vorrei ringraziare tutti voi senatori per la fiducia che mi avete accordato. Per me è un onore essere qui. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 951, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza

Signor Presidente, devo purtroppo riferire che la 1a Commissione, che presiedo, non ha potuto completare l'esame di questo importante disegno di legge di conversione per i tempi troppo limitati a nostra disposizione e per il numero, relativamente alto, degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati. Ieri sera, nella seduta delle ore 20, abbiamo dovuto prendere atto che atto che concretamente non c'era il tempo sufficiente per licenziare il provvedimento e votare il mandato al relatore entro questa mattina.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

Ha chiesto di intervenire la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

un fenomeno strutturale, quale quello delle migrazioni, in chiave e con strumenti di natura squisitamente emergenziale. È la quarta volta che dedicate a un decreto-legge ai migranti: la quarta. Disposizioni urgenti sono state anche quelle del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il cosiddetto decreto mezzogiorno e immigrazione, così anche il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che recava disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione marzo 2023, n. 20, che recava disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare così pure il decreto del 14 settembre 2023 del Ministro dell'interno, che indica l'importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero nel corso della procedura per accertarne il diritto di accesso in territorio nazionale. Quest'ultima è una previsione veramente ingiusta, Presidente, che è già stata disapplicata dai tribunali più volte, perché contrastante con la Costituzione e con la normativa comunitaria. i presupposti di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, sono presenti almeno stavolta? Io direi di no, assolutamente no. Il Governo, invece di affrontare la questione dell'immigrazione con iniziative organiche, in armonia con quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa europea, preferisce, anche con una produzione legislativa di qualità direi discutibile (tant'è vero che al vaglio della magistratura cade pietosamente), passare di emergenza in emergenza. Ce lo state dimostrando quotidianamente: il susseguirsi di decreti-legge ne è la conseguenza. Noi vi chiediamo di fermarvi. Questo decreto-legge è per noi incostituzionale, come lo erano i precedenti. Basta leggere l'articolo 5 che, al comma 1, alla lettera *a)*, prevede che, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee, il prefetto possa disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore ai sedici anni nelle strutture per adulti,

tanto più che il combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, prevede, in caso di estrema urgenza, cioè sempre, la deroga al limite di capienza fino al 50 per cento in più dei posti previsti, così determinando una situazione in cui i minorenni dovranno, in pratica, convivere con gli adulti. In quale situazione poi? In una situazione di promiscuità e affollamento estremo, in contrasto anche con il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Né vale l'utilizzo strumentale dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, che prevede la possibilità di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo se è nel loro interesse superiore. Questo perché, in questo caso, è evidente che ci si riferisca, ad esempio, all'ipotesi di un minore che non venga separato da un adulto di riferimento. L'articolo 5 di questo decreto viola anche la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, con la legge n. 176, in vigore tutt'oggi in 193 Stati, che prevede la collocazione di minori di età, privi di ambiente familiare, in adeguati istituti a loro dedicati. L'Italia, vi rammento, è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione dell'articolo 3 della CEDU, nel caso di un minore trattenuto in un centro per adulti a Como. La sentenza è del 31 agosto 2023. Devo ricordarvi anche che l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, esclude che il minore non accompagnato possa essere trattenuto o accolto presso i centri governativi? Questo decreto consente anche di accertare l'età del migrante non accompagnato, che si dichiari minore, mediante rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici. Questo non è accettabile. Già il famigerato decreto Cutro aveva eliminato l'assistenza psicologica, l'informazione legale e di orientamento per i migranti. Adesso, vi è questo nuovo decreto: ma fino a che punto vogliamo arrivare, signora Come se non bastasse, abbiamo anche la previsione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, che introduce un procedimento diretto a stanare, nell'intenzione del Governo, i maggiorenni che si fingerebbero minorenni. Ora, questa norma stabilisce un termine per impugnare che è di soli cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Io direi che è chiaro e palese il contrasto con le garanzie processuali e con il diritto alla difesa previsto e garantito a tutti dalla Costituzione, anche agli immigrati. Non mi soffermerò sulle nuove disposizioni sul gratuito patrocinio, anche queste in aperto contrasto con il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione. Insomma, per tutti questi motivi, vi chiedo di non procedere alla conversione in legge di questo decreto e di votare a favore delle questioni pregiudiziali.

lavoro. Io temo di essere estremamente pedante questa mattina, ma lo sono perché credo profondamente nel valore del potere legislativo del Parlamento. mi serve essere pedante e tornare anche al mio vecchio mestiere di professoressa. Io dubito, ma magari sarò smentita dai colleghi, che all'interno di quest'Aula tutti i colleghi siano a conoscenza di che cosa in giornata voteremo. Perché dico questo e per quale motivo noi abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP2? Al netto del fatto che non è ancora chiaro, e che non riuscite a spiegarcelo, dove sia la straordinaria necessità e urgenza che ha spinto alla realizzazione di questo decreto, ci troviamo di fronte ad un ennesimo decreto-legge, che arriva di corsa (in questo ramo del Parlamento è arrivato ieri,

per approfondire il provvedimento, studiarlo, presentare gli emendamenti ed essere pronti ad una discussione, immagino che siamo tutti preparati. Siccome ne dubito, perché mi sono messa a leggere il provvedimento e ci ho impiegato parecchio (anche perché contiene tutta una serie di riferimenti a provvedimenti precedenti), mi sono detta che forse questa mattina poteva essere il caso di spiegare, come farebbe una professoressa in classe, il perché delle motivazioni che ci portano a dire che per noi è necessaria una pregiudiziale pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, al fine di non procedere all'esame di quest'atto.

nel quale vengono introdotte alcune previsioni relative alla possibilità di accogliere in via provvisoria i minori ultrasedicenni nelle strutture di prima accoglienza e accoglienza straordinaria. Quali sono queste strutture? Non sono strutture per minorenni, ma per adulti. Tali disposizioni creano quindi un grave allarme sotto il profilo della promiscuità che verrebbe inevitabilmente a crearsi tra adulti e minori, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza del minore. *(Brusio)*.

dicevo, tali centri non sono adatti a garantire l'accesso dei minori e tolgono dei diritti fondamentali come il primo colloquio o l'accesso ad un'assistenza psicologica adeguata alla loro condizione di vulnerabilità.

fondamentale e al centro di tutta l'azione il rispetto del superiore interesse del minore. *(Applausi)*. Colleghi della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, dov'è in questo caso il rispetto del superiore interesse del minore? Tralascio il fatto che questa norma porta a una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri, in palese violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo *(Applausi)* e delle numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori.

dice che ci può essere la possibilità - e lo dico al Governo, che magari l'ha anche sottolineata - di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo se è nel loro interesse superiore, e cioè per non rompere il legame con uno degli adulti lì presenti, quindi per mantenere un legame familiare o un rapporto già costituito; solo in questo caso. *(Applausi)*. Lo dice - lo ripeto - una direttiva europea. andrei avanti, richiamando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio del 1991 con la legge n. 176, nella quale la collocazione dei minori di età privi di ambiente familiare debba essere fatta in adeguati istituti a loro dedicati e non opera alcuna distinzione nei confronti di chiunque abbia un'età inferiore ai diciotto ma riconosce il diritto di ciascun minore a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso da rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni né differenziazioni in base alla nazionalità,

Ma veniamo alla procedura introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che prevede che in caso di arrivi consistenti multipli e ravvicinati, l'Autorità di pubblica sicurezza possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti

che ha stabilito il protocollo multidisciplinare per la determinazione dei trattamenti da tenere nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e non è riscontrabile nessuna eccezione possibile da applicare in

2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati - che viene di fatto smantellata che declina punto per punto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che l'Italia ha recepito. Per smantellare una legge di iniziativa di una parlamentare del Partito Democratico, smantellate l'accordo e la Convenzione ONU, non so se ve ne siete resi conto.

La ringrazio. Signor Presidente, colleghe, colleghi, senatori e senatrici, componenti del Governo, capisco, capisco, dalla reazione alle questioni pregiudiziali poco fa presentate, che in questa Aula c'è uno scarsissimo interesse al nostro ruolo. C'è in realtà l'idea che non sia il Parlamento il luogo della legislazione - ruolo che ci affida la Costituzione, ma anche gli elettori quando ci eleggono in Senato e alla Camera - e ci sia invece l'idea che è meglio proteggersi, non aprire nessuna discussione, non provare ad avere dei livelli di confronto, forse perché altrimenti le scelte quotidiane di questo Governo metterebbero in difficoltà gli stessi rappresentanti della maggioranza. Eppure, come organo legislativo quale siamo, abbiamo in realtà l'obbligo di rispettare non solo la Costituzione del nostro Paese, non solo la legislazione, ma tutte quelle convenzioni e quei trattati internazionali che regolano innanzitutto la convivenza tra i Paesi e il rispetto delle regole. È stato già detto dalla collega Malpezzi che il decreto-legge che stiamo discutendo viola l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interviene e viola la direttiva n. 33 del 2013 dell'Unione europea. Non sono due fatti indifferenti.

forse la prima cosa che dovremmo fare è rispettare le convenzioni e le direttive, proprio per avere quell'ascolto che oggi diciamo di non avere. Vi abbiamo detto poco fa che basterebbero queste violazioni, oltre a quella dell'articolo 77 della Costituzione, per non procedere nella discussione sugli articoli 4 e 5 di questa legge. che la Camera ha peggiorato nelle sue previsioni, che presentano soprattutto un elemento. Possiamo infatti ripercorrere tutto quest'anno di legislatura una domanda alla fine comincia a emergere: ma che cosa ci hanno fatto i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine per dover subire un costante livello di odio e di pregiudizio? Che rapporto pensiamo di avere con le nuove generazioni, che siano stranieri o meno, se è sempre fondato sulla diffidenza, la repressione, una voglia di una normalità che viola innanzitutto il loro star bene e crescere? Devo dire che non ho trovato nessuna risposta a questa domanda e continuo a domandarmi, visto che abbiamo uno strano gusto che si ripete di decreto-legge in decreto-legge (come è stato ricordato, siamo al quarto decreto-legge nel giro di un anno sul tema delle migrazioni) se siamo coscienti, come senatori e senatrici e come onorevoli alla Camera, di essere un Paese sottoscrittore e quindi tenuto all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le previsioni che infatti sono determinate per i minori non accompagnati stranieri sono di pura violazione.

che i bambini potranno vivere in carcere con le loro madri, tornando indietro rispetto a tanti principi acquisiti. Vorrei quindi ragionare con voi su che significato ha per il Parlamento italiano non attuare il concetto di interesse superiore del minore come facciamo a confrontare le scelte legislative che questo Parlamento dovrà fare nelle prossime ore con la convenzione europea secondo la quale i minori possono essere collocati con adulti solo se è nel loro interesse superiore.

in merito al superiore interesse del minore non può prevaricare l'obbligo di rispettare i diritti del minore stesso. Guardate che all'interno di questo commentario c'è un principio fondamentale, quello per cui bisogna occuparsi del minore e non di che cosa l'adulto vorrebbe che il minore facesse. Ancora, innanzitutto perché così viene detto - esiste il diritto del minore di essere libero da ogni forma di violenza; anzi, abbiamo l'onere e l'onore della loro protezione. Vorrei quindi domandare a voi se la reclusione, di fatto per la sola colpa di essere arrivato nel nostro Paese, è una forma di violenza; se cambiare il protocollo rispetto al trovare e verificare la certezza dell'età di un minore è una forma di violenza, quando appare lasciata alla discrezionalità di chiunque venga incontrato da quel minore e non più accertata, come stabiliva la norma precedente. Ancora, dire che non si segue il protocollo multidisciplinare perché ci può essere l'urgenza, non è forse esattamente un'invasione della vita di quel minore e della sua, invece, necessaria protezione?

tenendone conto in qualunque procedimento decisionale; deve, inoltre, essere un diritto individuale che tenga conto delle condizioni di ciascun minorenne al fine di promuoverne e garantire il benessere in termini di bisogni primari, materiali, fisici, educativi, emozionali. Permettetemi allora di chiedervi, rispetto al decreto-legge in esame, alle norme che avete introdotto, allo smantellamento della normativa precedente, in che cosa rispondete al promuovere e garantire il benessere in termini di bisogni primari, materiali, fisici, educativi ed emozionali. Il colloquio, il supporto psicologico, lo studio, oltre che un luogo sicuro, non sono strumenti difficili da individuare, erano già tanta parte della nostra normativa.

Potrei continuare su molti degli articoli e delle caratteristiche del decreto-legge in esame; lo faranno poi, anche con maggiore autorevolezza, i colleghi che interverranno. Vorrei però riproporre la seguente domanda: perché volete imporre al Paese la cancellazione del superiore interesse del minore? Perché non volete rispettare la nostra Costituzione? Ricordo che in queste Aule lo urlavate voi, anche con toni ben diversi da quelli che usa l'opposizione in questa legislatura. Ora che siamo ormai in grado di poter dire e testimoniare che altri Governi hanno fatto un uso più limitato di voi dei decreti-legge, dell'estrema urgenza, della legislazione immediata e così via, vi domando quanto segue: se non volete ascoltare le nostre ragioni, le ragioni dell'opposizione, perché non provate ad ascoltare voi stessi?

quello che discutiamo è il quarto decreto-legge in un anno sul tema migranti ed è sempre lo stesso film, quello di norme in pericoloso attrito con il diritto internazionale, inasprimenti senza efficacia sul piano della deterrenza, ma che ogni volta segnano un sinistro arretramento sui principi di umanità e di tutela della dignità delle persone. Sull'immigrazione il Governo ha messo in moto una spirale propagandistica senza precedenti, che si frantuma in mille pezzi davanti ai numeri: 152.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, il 50 per cento in più rispetto al 2022, ennesima conferma che il modo con cui la destra affronta il tema migratorio non è la soluzione, ma è parte del problema. Sono più di vent'anni, da quella legge Bossi-Fini che introdusse il reato di immigrazione clandestina, che la destra vende all'opinione pubblica l'idea che la migrazione vada affrontata come una questione di ordine pubblico. Invece le migrazioni sono - ahinoi - un tema che richiederebbe ben altra postura. Le migrazioni ci parlano di cambiamento climatico e di riassetto degli equilibri geopolitici; interpellano l'Europa e la sua ragion d'essere dovrebbero porre una questione essenziale per un Paese che vive un drammatico inverno demografico. Oggi il più potente *pull factor* all'immigrazione non sono le ONG, come sostiene il ministro Piantedosi, ma ad esempio i negazionisti del clima. Se non si arresterà il cambiamento climatico, sulla direttrice Nord-Sud nei prossimi anni si metteranno in marcia milioni di persone. E non saranno certo gli accertamenti socio-sanitari sulla reale età dei migranti a convincerli a non partire. Ma non è solo questo. L'Africa vive una condizione di estrema instabilità: la Libia, il quasi *default* della Tunisia, l'Egitto, su cui si scaricano parte delle tensioni del conflitto tra Israele ed Hamas, il Sahel, dove negli ultimi anni si sono verificati tutta una serie di colpi di Stato militari. E poi le mire della Cina sui Paesi più ricchi di terre rare, le strozzature russe nelle forniture di grano per scatenare nuovi flussi migratori e tramutarli in un'arma di pressione politica sull'Europa. L'Africa e più in generale il Mediterraneo sono diventate il punto di caduta delle tensioni che attraversano il mondo, dimostrando che ciascuno di questi teatri appartiene a una crisi globale, che non si affronta in solitaria con un Piano Mattei dai contorni alquanto fumosi, che rischia di generare soltanto confusione tra la futura struttura di missione, il nostro corpo diplomatico e lo stesso Ministero degli esteri, ma che richiede un'Italia capofila all'interno delle sue storiche alleanze. Penso naturalmente all'Europa, con il superamento di Dublino, ma anche con quel protagonismo sulla scena globale che è clamorosamente mancato in questi mesi. E penso soprattutto alla NATO, attraverso un'azione di sensibilizzazione per il rafforzamento del fronte meridionale dell'Alleanza, che è quello ad oggi più trascurato e che invece richiede le stesse attenzioni destinate al fianco orientale o a quello dei *partner* dell'Indo-Pacifico, anche perché i punti di contatto e le connessioni con gli altri scenari sono molteplici. Il coinvolgimento dell'Europa e della NATO è essenziale per stabilizzare il Mediterraneo e l'Africa dalle potenziali minacce, non ultima quella per i nostri approvvigionamenti energetici, dopo che abbiamo giustamente sostituito Mosca con una serie di accordi siglati in Africa. Poi c'è un'altra questione: nel 2050 il mondo avrà 9,7 miliardi di abitanti. Quanto può contare un Paese che rischia di scendere a 54 milioni? Per invertire la tendenza non bastano le politiche per la famiglia, ma serve una politica delle quote migratorie che accolga e formi nuovi italiani secondo le regole dell'integrazione. Occorre allora rispolverare parole che sono state completamente rimosse dal nostro vocabolario pubblico: quote di ingressi, canali umanitari, *ius culturae*. Occorre cioè smettere di pensare all'immigrazione come a un problema di ordine pubblico o, peggio ancora, come a una forma di devianza sociale, per fare finalmente i conti con la realtà. È la tenuta sociale ed economica del nostro sistema pensionistico, ad esempio, è il ruolo che l'Italia vuole avere nel mondo a chiedercelo. Insomma, tutto serve, eccetto quello che sta facendo questo Governo, perché, anche a volerlo seguire nella strategia delle pene e degli inasprimenti, senza accordi per i rimpatri e senza il superamento di Dublino è soltanto una straordinaria messa in scena, una *fiction* girata sulla pelle di chi più soffre, con l'effetto non secondario di consegnare quote di disperati nelle mani dei caporali, degli sfruttatori della prostituzione e della criminalità organizzata. Vere e proprie bombe sociali piazzate nelle nostre città, in quei quartieri dove già è forte il malessere sociale, per alimentare l'equazione, sempre utile ai dividendi elettorali, dello straniero come minaccia per la collettività. Non è così che si guida un grande Paese. Non è così che lo si dota di una visione del futuro. Non è così che si trattano i principi di umanità, parte fondante della nostra storia, della nostra Repubblica e della nostra collocazione europea. E allora tornano alla mente le parole di un grande italiano: «i nostri confini, in alcuni casi, sono diventati confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità, muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra e dalla povertà»; «l'unica soluzione è una politica comune europea che salvaguardi il diritto d'asilo e regoli i flussi migratori». Quell'italiano era David Sassoli *(Applausi)*: se potete, fatene tesoro cominciate ad affrontare la questione per come merita e ad ascoltare le voci che anche nel vostro campo dicono che è il giunto il momento di governare l'immigrazione in un'ottica diversa,

Signor Presidente, mi consenta di farle le mie congratulazioni e di augurarle buon lavoro. Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'instabilità politica e sociale del continente africano, in particolar modo nel Sahel, contribuisce a un incremento del fenomeno migratorio verso l'Italia e l'Europa. Dalla fascia saheliana, infatti, si possono gestire e indirizzare gran parte delle migrazioni dirette verso l'Europa, a maggior ragione oggi che, se la notizia viene confermata, il Niger ha abrogato una legge del 2015 che considerava illegale il traffico dei migranti. È quindi innegabile che i paramilitari legati alla Russia presenti nell'area stiano incentivando le partenze, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i Paesi considerati ostili dal Cremlino. Nella zona sono inoltre in corso conflitti tribali, religiosi e politici, e negli ultimi anni si sono sviluppate importanti connessioni tra gruppi criminali e organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Diventa perciò oggettivo riconoscere che l'immigrazione irregolare può rappresentare una minaccia per la sicurezza della nostra Nazione e dell'Europa, a maggior ragione dopo i tragici fatti del 7 ottobre scorso in Medio Oriente. Il caso dell'autore dell'attentato del 16 ottobre a Bruxelles dimostra che sui barconi che arrivano sulle coste italiane si possono confondere anche soggetti radicalizzati, pronti a colpire nelle principali città europee noi, l'Occidente, le nostre radici, la nostra cultura e la nostra identità. In modo preventivo e lungimirante, quindi, il Governo italiano con questo decreto ha previsto importanti misure per aumentare la sicurezza sul nostro territorio e in materia d'immigrazione, come il divieto d'ingresso in Italia degli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesioni personali, fra cui voglio ricordare la mutilazione dei genitali considerata reato in Italia dal 2006, con la legge Consolo. Il decreto prevede inoltre espulsioni più rapide per motivi di ordine pubblico e sicurezza anche per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; prevede il contrasto al fenomeno delle domande reiterate presentate in modo pretestuoso e dilatorio mentre è in corso la procedura di rimpatrio e nuove regole che consentiranno di accertare celermente celermente l'età reale dei migranti minori non accompagnati, soprattutto nella fascia tra i sedici e i diciassette anni (che sono più del 70 per cento), al fine di offrire le tutele destinate ai fragili solo a chi ne ha veramente diritto e non a chi mente. A proposito di diritto non ho sentito dire nulla, ma grazie al Governo Meloni le tutele previste solo per le donne migranti in gravidanza e con minori sono state estese a tutte le donne, senza distinzioni. una misura di grande civiltà, cui nessun Governo aveva mai pensato prima. In questo modo, si riduce la possibilità di promiscuità nei centri e che le donne possano subire violenze o essere preda di sfruttatori della prostituzione, ma non solo. Il decreto prevede anche l'aumento di 400 unità del contingente Strade sicure da destinare alle principali stazioni ferroviarie italiane, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità di questi luoghi ai cittadini, ma anche ai turisti. inoltre il rafforzamento del contingente della Guardia costiera e vari stanziamenti fino al 2030 a favore di Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale flusso migratorio. In questo anno il Governo Meloni ha affrontato la questione dei migranti irregolari con una determinazione e un pragmatismo apprezzati anche in Europa, tanto che la stessa Ursula von der Leyen, quando è venuta a Lampedusa, ha usato le stesse parole del nostro Presidente per dire che non spetta agli scafisti decidere chi debba entrare in Europa *(Applausi)*; concetto che ha anche ribadito non più tardi di due giorni fa alla Conferenza per un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. Tutto ciò a dimostrazione di quanto sia cresciuta la credibilità dell'Italia in Europa grazie al lavoro del nostro Presidente del Consiglio. L'impegno degli altri Stati europei, da un lato, e la collaborazione con i Paesi africani, dall'altro, sono strategici per gestire la questione dei migranti irregolari. L'accordo con la Tunisia lo dimostra: da ottobre, per la prima volta dal 2022, si è registrato un calo degli arrivi di migranti La guardia costiera tunisina, dal 22 ottobre al 23 novembre, ha bloccato 63 operazioni di migrazione clandestina via mare, intercettando e salvando ben 1.267 persone, arrestando scafisti e sequestrando sequestrando barche. Questo è un chiaro segnale da parte della Tunisia di voler rispettare con serietà e fermezza gli accordi siglati con l'Italia. Voglio ricordare in questa sede anche il patto con l'Albania; un patto di portata storica che, in un momento di fortissima pressione migratoria, permette di alleggerire il carico sull'Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri. Un altro successo del nostro Presidente del Consiglio sul piano internazionale, che, assieme all'accordo con la Tunisia, rappresenta un modello replicabile di cooperazione tra Stati nella lotta al traffico di esseri umani e per la gestione dei flussi migratori in un quadro di legalità e a cui molti Stati europei stanno guardando con interesse e - io aggiungerei - anche con ammirazione. L'annuncio ha chiaramente colto di sorpresa la sinistra, che pensava che quest'estate Giorgia Meloni fosse andata in vacanza in Albania perché si spendeva meno che in Italia. Una sinistra che, come ha detto al *Premier question time* il presidente Meloni, non ci ha visto arrivare e che, non sapendo cosa dire pur di criticare a prescindere, è addirittura arrivata a paragonare i centri che verranno realizzati a luoghi di deportazione, come a voler insinuare che in Albania i diritti umani non vengono rispettati, offendendo il popolo albanese, dimenticando che l'Albania fa parte della NATO e del Consiglio d'Europa ed è candidata ad entrare nell'Unione europea. Ma a far loro notare lo scivolone (e uso un eufemismo) ci ha pensato lo stesso primo ministro Rama, per cui non mi dilungo. Il Governo Meloni, però, vuole fare di più. Vuole sradicare le motivazioni che spingono tanti africani a migrare. Il Piano Mattei va proprio in questa direzione, perché prevede un modello di cooperazione e di supporto reciproco con gli Stati africani. Noi - ma anche l'Europa - abbiamo bisogno degli Stati africani sia per affrontare la questione della migrazione irregolare, sia per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento al fine di continuare ad affrancarci dal monopolio del gas russo. Si tratta, fra l'altro, di una strategia lungimirante premiata anche dall'agenzia di *rating* Moody's. Gli Gli Stati africani hanno bisogno di noi per svilupparsi, per progredire e perché i cittadini africani non siano più costretti a migrare per necessità. Purtroppo, favorendo le cosiddette primavere arabe, l'Europa e l'Occidente, sbagliando, hanno lasciato campo libero a Cina e Russia. È quindi fondamentale fornire agli Stati africani una valida alternativa all'espansionismo russo e cinese, garantendo un nuovo sistema di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, istituendo una cooperazione che possa comprendere un aumento delle esportazioni e aumentare gli investimenti in istruzione, formazione professionale, ricerca e innovazione. Con il Governo Meloni non ci sarà più un'immigrazione incontrollata, al contrario: la priorità sarà stipulare accordi e creare le condizioni per permettere l'arrivo di immigrati regolari compatibili con le caratteristiche e le necessità del nostro tessuto sociale ed economico, evitando quanto fatto negli anni precedenti, ovvero un'accoglienza indiscriminata e ideologica, penalizzante non solo per l'Italia, ma anche per gli stessi immigrati, dovuta all'incapacità dei Governi precedenti di avere una visione strategica e lungimirante di un fenomeno di dimensioni mondiali. Il Governo Meloni, invece, una visione strategica ce l'ha. Non solo perché è un Governo politico, che prende decisioni e se ne assume le responsabilità; non solo perché è un Governo che banalmente segue dei criteri molto semplici, ossia l'interesse nazionale, il pragmatismo, il buon senso, che ormai è diventato merce rara; ma anche e soprattutto perché è un Governo che ha il coraggio di cercare soluzioni strutturali e non di facciata ai problemi della Nazione. Vede, Presidente, avviandomi alla conclusione, noi non siamo come quelli che volevano abolire la povertà con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Noi non siamo come quelli che volevano rimettere in moto l'economia col superbonus, senza pensare alle conseguenze, senza pensare che la povertà si combatte creando posti di lavoro e senza pensare che il superbonus avrebbe scassato le casse dello Stato. Ecco, noi non siamo così; noi vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi un'Italia migliore. Questo è l'impegno che ci siamo presi con gli italiani e su questa via proseguiremo.

gioia nel vederla sedere al banco della Presidenza: è un'ottima scelta che ho condiviso. Devo dire subito che sui diritti dei minori, impegno al quale ho dedicato tutta la mia vita, non faccio sconti a nessuno, né politici, né partitici. Fa parte della mia vita non difendere, ma occuparmi nel modo migliore dei minori. Secondo: rispetto all'immigrazione, la persona migliore deve arrossire, perché tutti noi siamo stati manchevoli, da qualsiasi punto di vista: la destra, la sinistra, palla al centro, sopra e sotto, tutti abbiamo mancato. Vedete, la migrazione di popoli nel lontano passato dal voler vedere cosa c'era oltre, oltre i confini: era un atto positivo. Gli uomini di Neanderthal hanno scoperto nuovi spazi, nuovi territori, nuovi modi di amare e di essere amati. Oggi è inutile che ci diciamo bugie: qualunque migrazione è figlia del dolore, il dolore per chi parte,

che ci ostiniamo indirettamente a difendere. Stiamo difendendo dei negrieri che sfruttano la vita di persone disperate. Ma ci rendiamo conto

ci mancherebbe altro, come l'aria, purtroppo troppo inquinata, anche qua dentro, da chi pensa che solo le sue idee siano quelle giuste e sono escrementi le idee degli altri. Ma ci rendiamo conto che danno psicologico, politico e umano creiamo in questo? Attacchiamo il Governo attuale di Giorgia Meloni perché tempestivamente cerca di dare risposte, a mio avviso ottime, anche se scomode in certi casi, e consideriamo questa tempestività voler chiedere consenso e pigliare in giro le persone. Quindi, se siamo tempestivi, sbagliamo. Se non interveniamo, come troppi Governi di grilli parlanti fanno in quest'Aula, pensando al non fatto precedente, insomma, questo doppiopesismo, per cui è meglio non fare nulla piuttosto che fare, mi sembra assolutamente tragicomico, se non ridicolo. Ma veniamo al punto,

dei quali in questi giorni abbiamo parlato, soprattutto delitti a carico di minori e di donne. Dobbiamo dire che non è giusto dire no a persone riprovevoli, veri e propri mostri? Come si fa a dire questo? Come si fa a dire: ma vengano pure coloro che provocano mutilazioni ai genitali femminili? Ma siamo tutti matti? Vogliamo inquinare anche i valori per i quali solo una settimana fa ci siamo battuti? Io provo veramente ribrezzo

certe volte, come ricchezza; troppe volte, creando uno stato di assedio. Dobbiamo dirlo, infatti: perché difendere solo l'immigrato e non chi vive e lavora da sempre nel nostro territorio? Questa cosa mi ha sempre provocato orrore, al di là della politica, al di là dei partiti. Ora parlo da tecnico. Sui minori, Sui minori, intanto stiamo parlando non di una penalizzazione teorica di tutti i minori non accompagnati. Tra l'altro, mi permetto di dire che, da Ministro della famiglia, nel 1994 cercai di potenziare tutte le azioni in favore dei minori non accompagnati. E proprio la sinistra mi impedì di fare di molto di più, perché dissero che facevo propaganda aiutando i minori non accompagnati. Provo ancora dolore per quell'accusa assolutamente sciocca, legata anche al traffico di organi. Mi presero per matto quando denunciai la cosa. Oggi se ne parla e si interviene a livello mondiale, riconoscendo che è uno dei pericoli più gravi dell'immigrazione non controllata. Ma torniamo ai minori.

parliamo di emergenza, parliamo di decisioni momentanee per salvaguardare le due fasce, anche con accertamenti, per vedere chi utilizza l'età in maniera impropria, per ottenere vantaggi impropri. di accertamenti seri, scientificamente provati, che sinceramente sono facili da gestire. Poi, per i minori inferiori di età, di luoghi assolutamente loro dedicati. In casi particolari, sarà il prefetto, che non credo sia un cretino, ma persona incapace di gestire i diritti dei minori, a gestire momentaneamente, nella prima fase, una possibilità di accoglienza dei minori accanto agli adulti, ma sempre in spazi dedicati e controllati. Se poi voi, perché non sono dei vostri, sfiducia totale nei prefetti, sfiducia totale nei tecnici che gestiscono i centri, allora andiamo tutti a casa. Infatti, nutrendo sfiducia

per chi impropriamente lascia il proprio Paese. Ha detto bene - sono abbastanza laico per poterlo dire - il Santo Padre: il diritto

Va rispettato il dolore di chi sta nella propria terra e si sente prevaricato, di chi deve lasciare la propria terra e si sente sradicato. dunque che la cosa migliore sia rispettare le scelte del Governo Meloni attuale, che quantomeno ci prova dopo anni di completo

non si preoccupi le daremo tutto il tempo.

non c'è nessuna necessità e urgenza, non c'è in particolare in questo caso e dirò subito perché. Il Parlamento viene umiliato per l'ennesima volta. Stiamo parlando di un decreto-legge che abbiamo a stento potuto leggere: lo abbiamo ricevuto ieri in Commissione; sono state date due ore per presentare degli emendamenti su un provvedimento di questo genere. Siamo in una situazione di monocameralismo di fatto.

dovrebbe farsi portatrice presso il Governo della difesa della dignità di questa Camera. Signora Presidente, le chiedo di voler informare il presidente La Russa perché credo che, soprattutto quando discutiamo di temi così importanti, avremmo il dovere, che la Carta costituzionale ci impone, di approfondire e di poter conoscere per poter deliberare. Qui, per definizione, si delibera senza conoscere. *(Applausi)*. Non c'è stato il tempo e trovo che questa circostanza vada denunciata chiaramente. Questa è la Costituzione vigente, noi abbiamo provato a cambiarla e purtroppo non ci siamo riusciti; forse sarebbe stato meglio. Detto questo, perché poi non possiamo considerare validi i requisiti di necessità di urgenza? Semplicemente per il fatto che qui non c'è nessun fenomeno straordinario. Il fenomeno migratorio è strutturale, come già altri colleghi hanno evidenziato, e dovrebbe essere affrontato in maniera strutturale. Il Governo cosa fa, invece? Questo credo che sia il quarto decreto-legge in tema migratorio e il Governo continua a sfornare norme che non danno una visione d'insieme e che soprattutto

al sottosegretario Molteni, eravamo colleghi, e devo dire che i Governi nei quali eravamo seduti insieme con la tanto vituperata ministra Lamorgese facevano risultati di gran lunga migliori di questo: l'anno scorso gli due anni fa erano un terzo degli attuali, a dimostrazione che le politiche di freno agli sbarchi non hanno nessuna efficacia. Ma soprattutto, la cosa che preoccupa è che il Governo continui a gestire questo come un fenomeno emergenziale, non rendendosi conto che abbiamo dei problemi strutturali. Signora Presidente, l'anno scorso sono nati 393.000 bambini; siamo scesi per la prima volta nella storia sotto i 400.000. In Calabria si è parlato di medici cubani, in Sicilia il Governo regionale ha appena aperto un bando per l'assunzione di medici stranieri. Viviamo un inverno demografico che già sappiamo ci metterà nelle condizioni di dover coprire posti di responsabilità con risorse umane, come si dice nel mondo aziendale, che l'Italia in questo momento non ha. Capisco benissimo che dobbiamo incentivare la natalità, ma per definizione la natalità è un progetto a lungo termine: concepire un medico oggi significa che quel medico sarà pronto ad andare in corsia tra trent'anni. Allora, la domanda che dobbiamo porre al Governo è come intenda riempire questi trent'anni, cioè come vogliamo gestire questo inverno demografico - l'Italia che invecchia - se non utilizzando la leva migratoria come fanno i Paesi più avanzati del mondo e come questo Governo non fa. Anzi, non solo non lo fa, ma prova a mettere in campo delle politiche che, tra l'altro, falliscono il più delle volte perché i suoi alleati in Europa impediscono che vadano in porto. La questione è semplicemente questa: in Italia non esiste un modo reale per immigrare in modo regolare. Quando ci si chiede perché i migranti arrivino sui barchini spendendo 8.000-10.000 euro, che sono costati il sangue delle loro famiglie, e con quei soldi non si comprino un biglietto per la *business class* per poter arrivare in aereo, la risposta è che non lo possono fare perché il biglietto di *business class* non è in vendita, non si può arrivare in Italia con un aereo, perché se si va a chiedere un visto ai nostri consolati, quelli non lo rilasciano. L'unico modo per arrivare qui, quindi, è appunto il barchino, affidandosi ai trafficanti, che poi vorremmo rincorrere intorno al globo terracqueo quando basterebbe tagliare loro

i nostri *click day* sono delle vere e proprie sanatorie mascherate, perché è chiaro che si tratta di lavoratori che stanno già in Italia, che poi magari devono andare a Lima a far finta di andarsi a prendere il visto in Perù, ma sono già qui, sono persone che conosciamo, che dovremmo regolarizzare subito, perché sono già in Italia, stanno già lavorando, stanno già curando i nostri anziani e le persone che hanno bisogno di cura. Noi invece le facciamo andare in Perù nella finzione che siano lì e che noi le abbiamo assunte lì, ma è ridicolo, perché sappiamo che di queste persone abbiamo bisogno. Quello che vorremmo sentire dal Governo è qual è il piano per far fronte a questo gelo

quindi degli italiani che sono all'estero e che non possono più rientrare, non nascono bambini, non facciamo un utilizzo intelligente del fenomeno migratorio e qual è la risposta del Governo? Arrivare qui con un decreto-legge trimestrale che va a stringere le maglie di un fenomeno che invece è vitale per il Paese. *(Applausi)*. Con tutto il rispetto e la stima per il senatore Guidi, quando ci parla di emergenze, nostro è il quinto Paese in Europa per richiedenti asilo. L'Austria, che ha meno di 9 milioni di abitanti, ha più richiedenti asilo dell'Italia e - udite, udite l'Austria non ha confini marittimi e confini esterni, perché confina con la Slovenia e con l'Italia, quindi i richiedenti asilo che arrivano in Austria sono movimenti secondari che in Austria non dovrebbero arrivare mai. Quando andiamo in Europa a parlare di emergenza,

Camera è stato difficile far accettare anche semplicemente l'educazione sentimentale nelle scuole per un senso di protezione dei bambini, e allora i bambini proteggeteli non mandandoli in galera con gli adulti perché questo state facendo con una leggerezza che, credetemi, cari colleghi, fa spavento.

dal senatore Scalfarotto che, secondo me, nel metodo e anche nel merito ha detto parole giuste, che dal mio punto di vista sono molto condivisibili. Come ha detto lui e ripeto io, questo è il quarto decreto-legge in un anno dedicato

So bene che quella che si sta determinando in questa legislatura non è una novità e che ci sono alle spalle anche una serie di precedenti molto indicativi. Non è la prima volta che l'attività parlamentare va avanti solo ed esclusivamente attraverso l'uso dei decreti-legge, è un problema antico che, anno dopo anno, peggiora sempre di più. Mi sento però di poter dire che con questo Governo abbiamo battuto qualunque *record* non fosse già stato immaginato nel corso degli anni passati. Andiamo al ritmo di una fiducia a settimana, come abbiamo detto

che essa possa addirittura essere codificata, come si pensa di fare con la riforma costituzionale. Questo però è un altro discorso che verrà naturalmente quando affronteremo la riforma. Torniamo invece al merito del decreto-legge. tratta del quarto decreto-legge in un anno dedicato ai migranti. Veramente un'ossessione, lo dico al Sottosegretario che conosce il mio pensiero in materia. Io non voglio fare esercizio di benaltrismo, però in questo caso viene davvero da dirlo; in un Paese come il nostro, con la situazione sociale che conosciamo, con i problemi ben noti dei mutui, degli affitti insostenibili, dei salari fermi da trent'anni, dell'assistenza locale ridotta a brandelli, dei costi altissimi dell'energia, delle materie prime, del dissesto idrogeologico, dell'inflazione, delle varie questioni, come le ultime di queste ore, legate al mercato tutelato e alle persone che non sanno come pagare le bollette, in una situazione così drammaticamente clamorosa, noi individuiamo

Mi rendo conto, signor Sottosegretario, che siete costretti a farlo, perché quando si passano tutti i mesi della campagna elettorale, annunciando le "magnifiche sorti e progressive", spiegando al Paese che si risolverà la crisi sociale, la crisi sociale, che invece poi si presenta in maniera ancora più acuta e le varie ricette che vengono presentate non trovano nessun tipo di riscontro, allora diventa facilissimo utilizzare la questione migratoria come arma di distrazione più efficace: si parla dei migranti per nascondere il fallimento sulle politiche sociali che si sta determinando nel corso di questi mesi.

non soltanto davvero molto contestabile anche dal punto di vista etico, ma anche molto sbagliata, molto grave e finanche completamente inutile questa scelta di realizzare i cosiddetti nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, di allungare i tempi di trattenimento, fingendo peraltro di ignorare che le rivolte, i morti, gli atti di autolesionismo, i suicidi, le quotidiane vessazioni, gli abusi,

Aggiungo - e su questo davvero mi sento di sottoscrivere alcuni interventi che ci sono stati in Aula stamattina, fra tutti quello del senatore Scalfarotto che anche io considero particolarmente gravi e in questo caso davvero non mi spavento ad utilizzare l'aggettivo «disumano», le scelte che sono state introdotte sulla questione specifica dei minorenni. È probabile che su questo ci sia davvero un'ossessione, perché dei minorenni abbiamo

da quei minori non accompagnati che paiono essere di almeno sedici anni e per i quali è disposto un trattamento insieme ai migranti adulti. Devo dire che a me ciò provoca qualche elemento di raggelamento del sangue, proprio per le vicende che sono state ricordate e anche per alcuni paragoni macabri e drammatici che hanno a che fare con la storia non soltanto di questo Paese degli ultimi anni.

che nelle situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori il prefetto possa ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, in totale spregio alla cosiddetta legge Zampa, al decreto legislativo n. 142 del 2015, al cosiddetto decreto-legge accoglienza, che aveva come principio base proprio l'idea che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto, oppure accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri e i centri governativi di prima accoglienza. Quella che era per l'appunto una misura di civiltà viene radicalmente e clamorosamente messa in discussione e modificata, a mio avviso in maniera molto sbagliata. Alla Camera, in Commissione, la maggioranza parlamentare è riuscita nell'impresa, che sembrava impossibile, di peggiorare il testo del Governo. Il testo era già pessimo, intendiamoci, ma la Commissione alla Camera è riuscita in questa impresa impossibile:

che peraltro conosciamo bene: utilizzare e immaginare la guerra tra poveri come possibile risposta mediatica a una serie di problemi del Paese. Francamente questo mi sembra un modo di governare

tali sofferenze e tali disagi si aggiungono peraltro ai disagi di persone che, come sappiamo, affrontano viaggi particolarmente drammatici e quindi arrivano nel nostro Paese in una condizione già profondamente vulnerabile. Stiamo parlando (non dimentichiamolo mai) di 23.500 minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio e, siccome i posti disponibili nel sistema di accoglienza (SAI) sono 6.150, la differenza è presto fatta. *(Applausi)*. Non capisco cosa vogliamo fare di tutte queste persone: chiuderle tutte all'interno dei CPR? È questa la soluzione che immagina il Governo? come se non bastasse, avete previsto una piena discrezionalità nell'incrementare la capienza delle strutture e dei centri di accoglienza dei migranti

degli accordi con Paesi come l'Albania, che avete fatto recentemente per esportare l'immigrazione; avremo modo di discuterne nel corso delle prossime settimane. Si tratta peraltro di un accordo fatto, anche in questo caso, lasciando il Parlamento in una condizione di assoluto silenzio. Non avete coinvolto il Parlamento, già questa cosa di per sé rappresenta un elemento di grande problematicità. Insomma, penso che siamo dinanzi alla solita cosa che abbiamo visto sin dall'inizio della legislatura: propaganda, propaganda e propaganda, ma nessun tentativo reale di affrontare i problemi e di guardare alla vicenda immigrazione come a una grande vicenda strutturale. Continuate a considerarla una questione di pura emergenza; penso che con questa linea e con questa idea non risolverete i problemi e non metterete il nostro Paese in una condizione migliore di quella in cui si trova ora.

Signora Presidente, le auguro anzitutto buon lavoro. Gentili colleghi, Governo, l'immigrazione è un problema che ci portiamo dietro almeno dagli anni Novanta e che difficilmente vedrà diminuire i flussi negli anni a venire. necessario adeguare le risposte a questo fenomeno in modo strutturale e non solo con delle misure di emergenza. soprattutto consapevoli che l'Italia, per la sua collocazione geografica e la sua conformazione orografica, rappresenta l'anello debole della catena europea. Gli arrivi ormai segnano presenze provenienti da tutto il mondo in via di sviluppo, non solo dai Paesi africani, ma anche da molte realtà del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Per dare risposta a decine di migliaia di persone che scappano da Paesi in guerra, in cui i diritti individuali sono compressi, o semplicemente da Paesi poveri serve un approccio diverso: adesso le risposte devono venire soprattutto dall'Unione europea. Non basta indicare il Paese di primo ingresso, ovvero fermare i migranti alle frontiere e mandarli indietro per stabilire chi sia responsabile della presa in carico e della gestione di coloro che hanno fatto ingresso nell'Unione europea. Serve una nuova politica europea sulle migrazioni e il tema riguarda l'Europa nel suo insieme, posto che, come hanno evidenziato le politiche del Regno Unito in tema, molti migranti intendono addirittura andare oltremanica, proprio perché lì spesso trovano amici oppure parenti. L'Italia deve quindi dare le proprie risposte e trovare anche le proprie soluzioni normative, il più possibile strutturali. Lo deve fare anche in attesa che l'Europa prenda atto del nuovo fenomeno migratorio, a partire dalla difesa delle frontiere europee, che sono frontiere di singoli Stati, ma anche i confini di un'Unione di Paesi europei. Questo decreto pone il controllo delle frontiere e il contrasto all'immigrazione clandestina come punti fondamentali e disegna un articolato preciso, innanzi tutto per collegare il fenomeno migratorio alla questione di sicurezza delle nostre città e dei nostri territori. Le norme che ora individuano le persone straniere cui non è consentito l'ingresso per ragioni giudiziarie o che devono essere espulse per motivi di pubblica sicurezza pongono limiti ben precisi. Vengono quindi potenziati i controlli sulle domande di protezione internazionale e migliorate talune procedure per concederla. Vengono poi introdotte disposizioni più puntuali per gestire il delicato tema dei minori non accompagnati, innanzi tutto perché spesso è difficile identificare il minorenne in assenza di documenti e sappiamo poi quanto sia delicato il confine della minore come la intendiamo noi in Italia, anche perché molto spesso in alcune zone del mondo alcuni minorenni non hanno fisici

Il tema dell'identificazione di chi chiede protezione in Italia dev'essere vagliato attentamente, perché ne consegue la sua eventuale vita futura in Italia. quindi con favore anche tutte le disposizioni che rafforzano il ruolo e aumentano le risorse a favore delle Forze dell'ordine e di coloro che in divisa sono sempre in prima linea per gestire il fenomeno migratorio. Per concludere, diamo il nostro pieno sostegno a queste norme puntuali sugli aspetti della migrazione legale, che punta ad inserire soggetti integrabili, perché è quello che ci chiedono le nostre comunità. Ora però l'Europa deve fare la sua parte e considerare una volta per tutte quello migratorio come un fenomeno europeo, perfezionando le proprie regole e rafforzando le istituzioni e i presidi già previsti. *(Applausi)*.

Lo dimostra il fatto che avete votato contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità ed emerge un elemento costante in questa politica che porta avanti il Governo: il Governo: la sistematica violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Usate il pretesto dei casi di straordinaria necessità ed urgenza per continuare ad affollare quest'Aula di decreti-legge. In questo caso addirittura ci avete dato poco più di ventiquattr'ore per concludere l'*iter* legislativo in Senato, mettendoci in estrema difficoltà nel fare il nostro lavoro: in questo caso non possiamo toccare palla e non possono toccare palla neppure i vostri parlamentari, i parlamentari della maggioranza. Ve lo abbiamo già detto? Sì, ve l'abbiamo detto, lo abbiamo detto milioni di volte, ma ve lo ripetiamo perché sembra che ancora non vogliate capirlo, che facciate finta di non volerlo capire. State continuando a calpestare la Costituzione. Diciamo pure che ci avete preso l'abitudine a calpestare la Costituzione perché, fondamentalmente, a voi la Costituzione non piace, è un fastidioso ostacolo. Cosa fare, allora, se non piace? O decidete di ignorarla, con un criterio di interpretazione giuridica creativa, oppure la cambiate. Avete immaginato adesso di introdurre un sistema folle di premierato, che non ha precedenti in nessun altro Paese del mondo. Costringerete i cittadini italiani a dare carta bianca a chi avrà fatto promesse elettorali e, se le tradirà, non ci sarà alcun modo di sfiduciarlo. *(Applausi)*. Mi viene da pensare l'esperienza di oggi ce lo conferma - che a voi non piace proprio la democrazia rappresentativa; volete non governare, ma semplicemente comandare e state sostituendo la democrazia con il pretesto di dover avere la possibilità di governare. La governabilità! Ci sono disposizioni in questo decreto-legge veramente aberranti. in particolar modo alle disposizioni che riguardano i bambini, gli adolescenti. Eravamo anche abituati a vedere un Governo che fa la voce grossa con i più deboli, ma quando si vanno a toccare i minorenni, se permettete, questa diventa una vigliaccheria istituzionale. istituzionale. Presidente, glielo dico da giurista: queste norme generano un sentimento che è di smarrimento giuridico. Qualunque giurista si rende conto che sono norme al di fuori di ogni contesto giuridico e culturale del nostro Paese. Si prova sconcerto. Ne hanno già parlato alcuni colleghi e se ne era parlato nelle due questioni pregiudiziali. Avete inventato - è questa l'aberrazione giuridica - una sorta di presunzione di maggiore età, attraverso queste misurazioni che trattano le persone come se fossero bestiame. Fate le misurazioni pensando che quelle siano adatte per stabilire se quel bambino abbia compiuto diciotto anni. Una presunzione che mi sembra anche contraria ai vostri principi di garantismo, a meno che voi non siate garantisti con i più forti e giustizialisti con i più deboli, perché questo mi sembra che sia l'atteggiamento del Governo.

E ancora - entrando sempre nel merito - state dimostrando l'amore per quel tipo di burocrazia che, piuttosto che avere il coraggio di dire un no, cerca di inserire un ingranaggio folle, che è la peggiore forma di diniego. Mi sto riferendo alla domanda di protezione internazionale. Abbiate il coraggio di dire che non vi piace la protezione internazionale, oppure non fate finta che tutto prosegua come prima, perché la state ostacolando attraverso un meccanismo burocratico, che andrà a penalizzare gli aventi diritto. Noi, come MoVimento 5 Stelle, Presidente, vogliamo essere custodi della democrazia, custodi dei valori della Costituzione e custodi dei valori della nostra società, che voi state purtroppo tradendo. parliamo dell'efficacia, perché voi siete andati al potere con la promessa elettorale di essere pronti a governare. Siete stati talmente pronti che state ancora rimaneggiando le vostre regole. Avete cominciato con un decreto sulle ONLUS, che non ha prodotto effetti;

ai vostri elettori - come li avevate già d'altra parte illusi in campagna elettorale - e avete visto che gli sbarchi sono aumentati. Anche quella misura è inefficace.

Allora, Presidente, qualche domanda ve la volete fare? Oppure pensate che si possa risolvere il problema dell'immigrazione con le stesse logiche fallimentari che avete adottato fino ad oggi? C'è bisogno di cambiare rotta. Cosa manca in tutti questi provvedimenti? Manca quello che normalmente un Governo dovrebbe fare per risolvere un problema del Paese, perché è come trovarsi su una nave che sta affondando e preoccuparsi di buttare via l'acqua a secchiate, senza pensare che bisogna anche riparare i motori, che bisogna riparare la falla. Manca la pianificazione. Non c'è nulla su cosa potrà succedere nei prossimi anni e non soltanto in questa legislatura. Non c'è nulla sulla cooperazione internazionale, che non si fa con il Piano Mattei, che non porterà ricchezza in nessuno di questi Paesi. In questi Paesi servono scuole, serve garantire il diritto all'istruzione e il diritto alla salute e servono iniziative dello Stato italiano italiano indirizzate verso una diplomazia che sappia contrastare le guerre, perché non ci dimentichiamo che la gente scappa dalle guerre, scappa da situazioni in cui si rischia di morire per la puntura di una zanzara e non ci si può curare. Scappano perché non si sa come dare un futuro ai figli, se non ci sono le scuole. Non c'è nulla in questo provvedimento, sempre messo in piedi sulla fretta istituzionale e su questa corsa, che poi vi costringe a un continuo rimaneggiamento e correzione di quello che avete precedentemente fatto.

Bisogna bilanciare la sicurezza con questo rispetto. Non può la sicurezza diventare il pretesto per calpestarli e voi state calpestando i diritti umani dei migranti e soprattutto dei minori. Questo francamente, Presidente, mi fa inorridire, ma quello che mi fa ancora più inorridire è la narrazione e l'uso del linguaggio, questa retorica anti-migranti, questa retorica che vuole alimentare la paura del diverso, questa paura atavica che forse può rafforzare il potere; la paura che il diverso sia sempre e comunque un pericolo. una narrazione che fa trattare i migranti e li fa definire come un carico residuale, come persone su cui si fanno delle misurazioni antropometriche. Ma vi rendete conto che qui c'è un problema

Però, vedete, io vi parlo dei diritti umani, ma non ne parlo solo io, non ve ne sta parlando soltanto il MoVimento 5 Stelle. Un articolo del «Corriere della Sera» di due giorni fa titola: «Minori migranti detenuti illegalmente»: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per l'*hotspot* di Taranto. Una notizia per un fatto datato, d'accordo, ma che contiene dei principi. È un

noi non possiamo che prendere le distanze da questo tipo di politica. Anzi, signora Presidente, forse è anche meglio che non ci abbiate dato la possibilità di emendare questo provvedimento, perché questo provvedimento non ha bisogno

vi sia la possibilità, da parte di un Governo, di portare in Consiglio dei ministri un provvedimento che vada contro le regole della Costituzione.

per esperienza politica ed amministrativa, che questo possa accadere. Quindi, si possono presentare le questioni pregiudiziali, si possono avere delle idee, ma la tesi che introduciamo regole contro la Costituzione e che sono disumane non rispetta i criteri delle istituzioni del nostro Paese.

In secondo luogo, con questo provvedimento, noi cerchiamo di dare una risposta ai tanti sindaci che sono in difficoltà, molti dei quali anche di colori politici diversi dai nostri. Sindaci che hanno già il problema dei minori nelle comunità, minori italiani, e che rischiano di averne anche di più con la presenza dei minori stranieri. Presidente, chiedo se è possibile parlare, oppure se c'è qualcosa che non va.

Non siete voi che potete dire quello che posso o non posso dichiarare durante la discussione generale. Stavo dicendo che il provvedimento cerca di rispondere alle esigenze di tantissimi amministratori, i quali chiaramente vorrebbero

difficoltà sulla gestione e l'applicazione dell'affido familiare, sui tutori legali. Ci sono tantissime difficoltà e quindi il Governo è intervenuto per cercare di trovare una soluzione. aspetti di disumanità, ma aspetti di gestione corretta per venire incontro ai nostri amministratori locali, che sono quelli che su queste tematiche soffrono tremendamente, perché questo Governo ha avuto il coraggio di ascoltare il loro grido di allarme.

l'hanno sempre voluta i capitalisti: lo scriveva un certo Karl Marx nel 1870 a proposito della questione irlandese. *(Applausi)*.

Il metodo in questo caso è anche sostanza e questo mi permette anche di rispondere indirettamente, signora Presidente, al presidente Romeo. Il problema di metodo è che continuare a porre fiducie su fiducie su questioni che riguardano

personali e fatti penali è un segno di debolezza da parte vostra, oltre che di mancato rispetto delle prerogative del Parlamento. *(Applausi)*. Penso che non ci sia la possibilità - lo dico ai colleghi di maggioranza - di fare dei confronti. Avete detto più volte in quest'Aula che siete una maggioranza politica, che disponete di un'ampia maggioranza politica. Un conto è porre la fiducia quando si ha un voto di vantaggio, ma con ampie maggioranze politiche e con l'opposizione che non ha intenzione di fare ostruzionismo perché non dibattere, se questo era il problema,

Con una maggioranza così ampia avete paura di non avere i voti? Quindi il decreto-legge già è uno strumento sbagliato. La seconda questione è la seguente: porre la fiducia continuamente con una maggioranza politica è un segno di grande debolezza, oltre che di mancanza di rispetto del Parlamento *(Applausi)*, e non facciamo confronti con altre maggioranze su questo

perché questo è uno degli elementi più importanti che dobbiamo mettere in campo quando parliamo del problema migratorio, sapendo che nessuno di noi ha la ricetta magica. Noi abbiamo fatto decreti-legge sull'accoglienza dei minori nel 2015 e nel 2017; abbiamo fatto una legge che riteniamo organica e molto valida; abbiamo fatto numerosi interventi abbiamo fatto numerosi interventi con il Ministro dell'interno, a suo tempo, per potenziare alcune questioni burocratiche e per semplificarle, ma nessuno di noi ha la ricetta magica. Non stiamo quindi facendo lezione al Governo, ma stiamo dicendo che la concretezza avrebbe richiesto, ad esempio, di considerare alcune questioni molto importanti. La prima è che siamo in presenza di una quantità di arrivi fuori misura, oltre i *record* precedentemente stabiliti anche da noi; siamo in presenza di flussi migratori totalmente fuori controllo. Guardo con grande simpatia alle dichiarazioni della collega di Fratelli d'Italia, che prima ci parlava di ben due accordi storici, ormai è tutto storico quello che fa questo Governo, forse sarebbe bene che si occupasse dell'ordinario, la storia la facciamo anche in altri momenti. *(Applausi)*. Ebbene, fra questi due accordi storici, prendiamo quello con l'Albania. Intanto, diciamo al Paese, signora Presidente, che ancora nessun migrante sta in Albania,

dell'ordine giuridico internazionale e ci saranno da chiarire numerosi problemi interni al Parlamento albanese, perché mi pare che il presidente del Consiglio albanese Edi Rama abbia detto al suo Parlamento che non saranno più di 3.000 i migranti che verranno

questo è un elemento su cui tutti insieme dobbiamo darci una mano, perché se la risposta è il Piano Mattei, che consiste nell'istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi, rimango un po' allibito a sentirla definire concretezza. Se il Piano Mattei è questo, allora siamo Vogliamo parlare di una cosa concreta? Parliamo delle file davanti alle questure per il rinnovo del permesso di soggiorno. *(Applausi)*. È dignitoso che un Paese civile continui a sottoporre a procedure burocratiche infinite persone che lavorano qui, che sono già qui da tempo, che non hanno nessun precedente penale, semplicemente perché non siamo in grado di mettere in piedi un sistema informatico di esame delle domande? Parliamo di cose concrete, parliamo del fatto che per la richiesta di protezione internazionale non bastano due anni, le commissioni territoriali e questo è un problema di diritto, certamente, perché nessuno vuole che rimangano qui persone che non ne hanno diritto. Nessuno di noi vuole che l'immigrazione venga decisa dagli scafisti, ma se vogliamo guardare in faccia la realtà, le risposte concrete che ci aspettavamo non erano sul piano penale, ma erano sul piano dell'esame più veloce, del potenziamento delle commissioni territoriali. Se vogliamo parlare del problema concreto, anzi concretissimo dei Comuni sottoposti a questa fortissima pressione migratoria, allora dovevamo parlare in maniera più forte dell'aumento dei posti nel sistema di accoglienza, dell'aumento e del coinvolgimento maggiore dei Comuni nel sistema SPRAR. *(Applausi)*. Sappiamo - l'ha detto molto bene il senatore De

che voi facciate queste cose per torturare i bambini, ma sto parlando di concretezza. Se ci sono 25.000 ragazzi minori sul territorio italiano e i Comuni sono 8.000, facciamo una divisione

bisogna andare incontro ai Comuni e bisogna mettere le prefetture nelle condizioni di istituire i centri di prima accoglienza per i minori. Non penso sia un problema insormontabile, ma allora perché non invitiamo i Comuni ad aderire al SAI

non alla velocità o all'arbitrarietà con cui un questore decide su una procedura. Pensiamo anche che le condanne che abbiamo ricevuto

Ho concluso, Presidente. Una legge che veda nel problema migratorio, come è stato detto da tanti miei colleghi, un problema strutturale e serio, ma anche una grande opportunità.

in maniera efficace dal Cardinal Parolin nella sua lettura magistrale alla Camera, come un problema strutturale che va affrontato con politiche interculturali, di rispetto, di convivenza e di assunzione dei valori più importanti della nostra convivenza

qualche timido segnale. Si può fare molto di più, si possono trovare le procedure anche in esperienze di altri Paesi moderni, come il Canada o l'Australia, dove le procedure di immigrazione sono semplici, ma garantiscono i veri diritti delle persone, senza trattarle come un pericolo. Non bisogna avere paura dello straniero se viene qui per lavorare, per mantenere la sua famiglia e per rispettare le nostre leggi. Non è uno straniero, è un cittadino come noi. Sono stranieri quelli che delinquono, che siano italiani da altri Paesi, non quelli che rispettano le leggi e vengono qui per mantenere la loro famiglia, come hanno fatto i nostri nonni per tantissimi anni quando in Italia non c'erano le possibilità che ci sono oggi.

Abbiamo ascoltato infatti un'unica discussione incentrata sul tema dei minori. Da questo decreto-legge però, che deve essere visto all'interno delle politiche sull'immigrazione di questo Governo e di questa maggioranza, bisogna trarne alcuni spunti, mettendone in evidenza altri che non sono stati trattati. provvedimento si inserisce in una politica del Governo che tende a dimostrare che l'Italia non è il Paese dove è importante entrare in qualsiasi modo, specialmente illegalmente, tanto poi dall'Italia non si esce più. Questo concetto è ribaltato dalla politica del Governo,

con le varie discussioni con i capi di Stato, africani e non, con il Piano Mattei e anche con quegli accordi che è giusto definire storici perché, non essendo mai stati fatti, sono innovativi rispetto al passato. Quello con l'Albania, che sappiamo dare molto fastidio perché nessuno ci aveva mai pensato, non è un accordo banale, perché si inserisce proprio in questo cambio di filosofia in questo cambio di filosofia teso a dimostrare a tutti gli irregolari che continuano ad arrivare sul nostro territorio, ma soprattutto a quelli che stanno pensando di arrivarci, che non basta più mettere piede a Lampedusa o in un altro *hotspot* italiano per avere la certezza di rimanerci vita natural durante, con o senza permesso di soggiorno, con o senza *status* di rifugiato. Anzi, questa certezza diventava assoluta quando si usciva dal circuito; diventava assoluta per tutti coloro a cui in cui veniva negato lo *status* di rifugiato o scappavano o non si presentavano ai posti di polizia quando dovevano declinare le loro generalità per mandare avanti la loro pratica, sia

i propri averi economici per essere poi mandato in un *hotspot* in Albania, che non è territorio italiano e da cui, se si esce, si è in uno Stato che non è l'Italia?

Pensate che il fatto che si arrivi in centinaia di migliaia, e che quindi non si può controllare chi arriva, possa essere messo a base del poter rimanere sul territorio nazionale? Noi pensiamo di no ed è per questo che il decreto-legge in esame si inserisce in un contesto maggiore di cambio di filosofia sull'immigrazione. Mi spiace che si sia posta tutta l'attenzione sui minori e desidero ribadire a chi definito giurista - e io non ho nessun problema ad ammettere che lo sia - che bisogna anche dire che le misure antropometriche per decidere se una persona è minore o meno non sono state introdotte dal presente decreto-legge, ma sono figlie della cosiddetta legge Zampa del 2017. Pertanto non è questo Governo inumano o contrario ai minori ad affermare che se non c'è altro metodo o altro modo per provare l'identità di una persona che si dichiara minorenne, se ne misurano

delle tutele destinate ai fragili e l'inserimento nel circuito della seconda accoglienza è per tutte le donne e non solo per quelle in gravidanza. Si tratta di un provvedimento di grande civiltà

Perché non dirlo, proprio nel momento in cui, a pochi giorni dal 25 novembre, queste norme vanno a favore delle donne, non solo di quelle incinte, ma di Perché non dire che finalmente c'è una norma che impedisce a monte l'ingresso in Italia di chi si è reso colpevole delle mutilazioni genitali, che è uno dei reati più schifosi che può essere compiuto verso le donne, o di tutti quegli uomini che all'estero hanno provocato lo sfregio per rendere irriconoscibile il viso delle donne? Perché non si può essere moralmente onesti e affermare che in questo decreto, a parte le cose che non vi piacciono, ci sono anche cose che per forza vi devono piacere?

di proporre provvedimenti che andrebbero contro la Costituzione. Il MoVimento 5 Stelle, attraverso di lei, Presidente, ha detto che i nostri provvedimenti non seguono l'etica italiana e qualcuno ha addirittura detto che noi siamo ossessionati dai migranti. La verità è che gli italiani sono ossessionati da quella parte di migranti che non vengono in Italia per studiare o per lavorare, ma vengono per delinquere e alimentano la microcriminalità nelle nostre periferie e non solo. *(Applausi)*. tutti benissimo che oggi la microcriminalità è nel centro delle nostre città, è nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi frequentati da giovani e non giovani. Se abbiamo, dobbiamo avere e crediamo nel rispetto per i minori stranieri, dobbiamo avere anche rispetto per i nostri minori tenendoli al riparo da certa criminalità che per la maggior parte è fatta da quella piccola parte di criminali stranieri che vengono in Italia per delinquere. *(Applausi)*. Per tutto questo noi siamo orgogliosi di questo provvedimento, che è stato che è stato già approvato dalla Camera con alcune modifiche significative, importanti e positive, e che oggi sarà approvato dal Senato della Repubblica.

Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. È convocata la Conferenza dei Capigruppo

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge immigrazione e sicurezza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, con inizio alle ore 14. Seguirà la chiama. Il calendario dei lavori della prossima settimana è integrato con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sull'oblio oncologico. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito i termini per la presentazione degli emendamenti ai decreti-legge previsti dal calendario. Gli emendamenti al decreto-legge prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei dovranno essere presentati un'ora dopo il termine stabilito per gli emendamenti in Commissione. Il termine di presentazione degli emendamenti al decreto-legge cosiddetto anticipi sarà fissato un'ora dopo la trasmissione ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione. È stato inoltre stabilito che mercoledì 13 dicembre, con inizio alle 9,30, avrà luogo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023. La consegna del testo delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati avrà luogo nel corso della seduta di martedì 12 dicembre.

il Governo di centrodestra si è posto l'ambizioso obiettivo di affrontare i problemi nazionali e internazionali con serietà e lucidità e la conseguenza è che il nostro *Premier* risulta, per questo, il politico più influente d'Europa, per coerenza e schiena dritta, che non le fanno difetto. *Ergo*, in merito al provvedimento in questione, i nostri sforzi sono stati a maggior ragione focalizzati sulla ricerca, non facile, di soluzioni in grado di governare il fenomeno migratorio e non solo di cavalcare quell'onda emotiva che troppo spesso tenta di dividere i buoni dai cattivi, alimentando l'innalzarsi di steccati ideologici e di tifoseria politica, distorcendo purtroppo la realtà dei fatti. In ballo non c'è solo il futuro del nostro Paese, ma c'è anche quello dell'Europa intera e delle risorse umane, economiche e di visione che sapremo mettere in campo. Il decreto-legge in esame arriva dopo l'eccezionale afflusso di migranti del 2023, con le conseguenze che inevitabilmente ne sono derivate sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mi preme premettere che il Governo ha sempre avuto come stella polare quella di provare a tutelare innanzitutto le vite dei migranti, cercando di combattere con tutte le forze il vergognoso traffico illecito di vite umane: uomini e donne che, con tutto il loro carico di speranze e di fiducia nei loro carnefici, troppe volte non arrivano nemmeno a sbarcare nel nostro Paese e diventa non un ponte verso la libertà, ma troppo spesso il loro cimitero. Il Governo Meloni, dunque, si è trovato a dover gestire, fin dall'inizio della legislatura, una vera e propria emergenza, peraltro sospettosamente anomala. E lo ha fatto seguendo le linee del programma, intervenendo sul fronte della politica estera e di raccordo con i Paesi dell'Unione europea, affrontando il fenomeno migratorio in senso strutturale, per tentare di eliminare alla radice la causa della pressione migratoria. Con un approccio di ricerca della complicità e di coinvolgimento, anche emotivo, delle istituzioni europee, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta giocando sullo scacchiere internazionale un ritrovato ruolo da protagonista dell'Italia; sta creando una sinergia inimmaginabile precedentemente con l'Unione europea; sta trattando singolarmente con gli Stati africani e con gli alleati al fine di costruire una fitta rete di relazioni che possano aiutarci ad affrontare seriamente il problema migratorio. Cito, ad esempio, la trattativa per la riforma del nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo o il *memorandum* europeo con la Tunisia del 16 luglio scorso, come pure il recente Accordo tra Italia e Albania in materia di immigrazione, che ha mostrato chiaramente la postura che questo Governo e questa maggioranza hanno inteso assumere di fronte al problema dell'immigrazione, ovvero fornire risposte sistemiche a una problematica strutturale che non faccia dell'Italia il campo profughi dell'Europa. Nessuno prima di noi aveva fatto tanto per la regolamentazione dell'immigrazione e coloro che, presi in contropiede, gridano allo scandalo, perché le soluzioni chiudono la bocca, sappiano che la Germania, l'Austria e la Francia stanno seguendo l'esempio italiano di *hotspot* fuori dall'Europa, che in fondo sono in linea con la mia proposta di isola artificiale europea, da più sbeffeggiata, nel Mediterraneo, per accogliere chi ha diritto a rimanere e rimandare nei propri Paesi i clandestini. A questo proposito esorto il Governo a utilizzare anche l'isola privata da 60 milioni di euro a Dubai che il narcotrafficante Quello che voteremo oggi sarà un'ulteriore provvedimento dedicato completamente all'immigrazione, dopo il decreto ONG e il decreto Cutro, a cui hanno fatto seguito gli altri importanti interventi sul territorio di Lampedusa e Linosa, approvati con il decreto Sud e il Piano Mattei. Le reazioni dell'opposizione, che ha paragonato le iniziative del Governo addirittura a una nuova Guantanamo o a un confino, sono state condannate dallo stesso *leader* socialista d'Albania, Edi Rama, che si è vergognato di essere estrazione della sinistra, ma anche - come detto sopra - dagli altri Paesi europei. accordi, peraltro, ci hanno permesso di registrare un sensibile calo degli sbarchi nei mesi di ottobre e novembre rispetto ai mesi precedenti, perché anche la prevenzione aiuta. Ebbene sì, la rotta dalla Tunisia ha segnato un netto crollo, a meno di non voler contestare anche le affermazioni della Commissaria europea degli affari interni Johansson, che ha dichiarato che c'è stato un calo dell'80-90 per cento dopo la sottoscrizione dell'accordo tra Unione europea e Tunisia. Per anni in quest'Aula ci siamo sentiti ripetere dalle sinistre che, se avessimo concesso la cittadinanza a tutti gli immigrati, essa sarebbe stata motivo di integrazione; che se avessimo introdotto lo *ius soli* nel nostro Paese, esso sarebbe stato un viatico per i futuri cittadini italiani per rispettare la nostra cultura, le nostre leggi, nonché motivo d'orgoglio e senso di appartenenza al nostro Paese. Per anni ci siamo sentiti ripetere che la soluzione per un'integrazione effettiva era l'accoglienza diffusa e distribuita tra i piccoli Comuni, perché - si diceva - è normale che nelle grandi città, in assenza di luoghi di aggregazione e in presenza di maggiori rischi di ghettizzazione periferica, gli immigrati fatichino a integrarsi. Forse, però, costoro non si sono accorti di una cosa: ci sono interi quartieri delle nostre periferie, nelle nostre città, che sono diventati invivibili; interi quartieri dove la tanto decantata integrazione è miseramente fallita dietro le decisioni, anzi, sotto le decisioni dei Governi con targa a sinistra. Persino nella mia città, che secondo tutti gli *standard* è la migliore in cui vivere, Bolzano, in realtà siamo ormai a un'involuzione sociale. Capiamo bene perché l'attività intensa e costante di questo Governo sul tema immigrazione sta facendo venire all'opposizione all'opposizione una crisi di nervi: per anni hanno subìto - e dico volutamente - un fenomeno che noi oggi governiamo e quello che proprio non riesce ad accettare è che ci stiamo riuscendo. Ci vuole tempo innanzi a decenni di lassismo, ma ci stiamo riuscendo. Continuano a ripeterci che l'emergenza non c'è, mentre i loro sindaci ripetono che l'emergenza c'è; i loro governatori dicono di no. I loro amministratori locali dicono di sì. Capisco voler fare opposizione, ma farla anche a se stessi mi pare francamente un po' troppo. La verità è che l'emergenza immigrazione c'è, cari colleghi, e noi la stiamo doverosamente affrontando, anche perché i cittadini italiani che pagano le tasse hanno diritto a vivere nel decoro e nella sicurezza. Quanto ai minori non accompagnati, nel 2022 sono scomparsi più di 13.000 minori stranieri dall'Italia, quasi il doppio dell'anno precedente. Rappresentano oltre il 75 per cento dei giovani di cui si perdono le tracce in Italia, e, per la stragrande maggioranza, hanno tra i quindici e i diciassette anni. Se quasi il 75 per cento dei minori italiani spariti viene ritrovato, per gli stranieri non si arriva nemmeno al 30 per cento. Nella migliore delle ipotesi, quei ragazzi sono riusciti a proseguire clandestinamente il loro viaggio. Al contrario, le ipotesi peggiori sul loro destino sono molte, troppe, agghiaccianti: accattonaggio, droga, pedofilia, prostituzione, traffico di organi. Le maglie delle reti criminali in cui possono finire questi questi ragazzi non lasciano molte possibilità di scampo. Abbiamo ancora la presunzione di pensare, sentendo questi dati, che avvolgerli in una coperta al loro arrivo sia sufficiente, magari con un panino e una bottiglietta d'acqua? Noi dobbiamo riservare adeguate tutele ai minori, a chi davvero ne ha diritto. Non basta farli entrare in Italia, se poi dobbiamo guardarli finire di nuovo, ancora una volta, nelle mani della criminalità, prima ancora che dei trafficanti di esseri umani. Se abbiamo il dovere di accogliere chi scappa da guerre, da carestie, chi fugge insieme ai propri figli o chi li lascia partire da soli, nella speranza di offrire loro un futuro migliore, abbiamo, allo stesso tempo, il dovere di decidere chi entra in Italia e quindi chi entra, di fatto, in Europa. Questo compito è delle istituzioni italiane e non possiamo delegarlo a scafisti privi di scrupoli. Il ritorno alla legalità, all'ordine sociale è la principale richiesta che il popolo italiano ci ha fatto con il suo voto. Questo decreto interviene per arginare proprio i problemi di legalità e sicurezza persistenti in alcune aree del nostro Paese e per evitare una *escalation* futura come quella cui abbiamo purtroppo assistito attoniti in Francia: sintesi, quindi, procedure più rapide per le espulsioni degli irregolari e dei migranti pericolosi, tutela dei minori veri, non di quelli finti, allungamento dei tempi di trattenimento nei centri di accoglienza, ma con priorità di riguardo verso le donne che giungono da noi e, soprattutto, rinforzo degli organici delle Forze dell'ordine. Negare oggi la fiducia al Governo, amici delle sinistre, significa dunque negare la fiducia alle nostre Forze dell'ordine, di tutti gli italiani, che sono in prima linea ogni giorno per contenere gli effetti della criminalità crescente, anche e soprattutto dovuta alla presenza di immigrati irregolari, ai tanti operatori del terzo settore, alla Croce Rossa internazionale, a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per debellare questa piaga. Come si può essere contrari alla rapida espulsione di soggetti ritenuti dediti a traffici delittuosi o che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica e morale dei minorenni, che offendono la sanità, che mettono in dubbio la sicurezza, la tranquillità pubblica? Come si può essere contrari alla più rapida espulsione di soggetti indiziati di reati di particolari gravità come il terrorismo? Noi la pensiamo come i cittadini. Siamo sempre dalla parte degli italiani e quindi daremo convintamente la fiducia al *premier* Meloni, al Governo e al sistema Italia. Concludo questa mia dichiarazione di voto, signor Presidente, con un ringraziamento particolare al ministro Piantedosi, al sottosegretario Molteni e al Ministero dell'interno per il lavoro quotidiano portato avanti nel contrasto all'immigrazione irregolare, per la sicurezza nelle nostre città e ai nostri confini. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo che presiedo, ripeto che continueremo convintamente a sostenere questo principio: in Italia si entra solo legalmente. Non arretreremo di un millimetro. Andremo avanti, perché vogliamo un'Italia più sicura, vicina ai propri territori, alle famiglie, alle imprese; perché vogliamo continuare a garantire legalità, certezza del diritto, attenzione ai più fragili e vulnerabili, come pure una sempre maggiore integrazione, ma solo per chi arriva legalmente nel nostro Paese. Stare a destra, nel centrodestra, come nell'accezione inglese *right*, significa stare dalla parte giusta, dalla parte del diritto. il testo di decreto-legge che ci accingiamo a discutere, sul quale poi è stato annunciato e richiesto dal Governo il voto di fiducia, è il terzo provvedimento d'urgenza con il quale il Governo

correttivi, principi, misure, in questo caso nuovi reati, nuove sanzioni, addirittura nuovi istituti, quale l'espulsione al posto della sanzione, per il soggetto che viene riconosciuto colpevole di avere dichiarato l'età falsa. di una serie di misure e di provvedimenti tutti introdotti con un decreto-legge. Noi non possiamo accettare e continuare a subire questa forma di decretazione continua da parte del Governo; una forma di decretazione che non è accettata, non è condivisa, neanche dal Presidente della Repubblica, che ha richiamato più volte il Governo sull'utilizzo corretto degli strumenti della legiferazione. legiferazione. Non è soltanto un modo artificioso attraverso il quale, invece di far legiferare entrambe le Camere, si ricorre a una forma parlamentare con una sola Camera che legifera, ma addirittura retrocede il ruolo della seconda Camera, in questo caso del Senato, a un mero organo ratificante. Questo provvedimento è stato trasmesso

un'ora e mezza per presentare gli emendamenti, con la consapevolezza che, dovendo il testo essere convertito in legge entro il 4 dicembre, cioè il in ogni caso non ci sarebbe stato il tempo neanche per esaminare quegli emendamenti, per dibatterli e spiegarli, per stimolare un confronto tra di noi. tutte le opposizioni hanno presentato degli emendamenti perché ognuno cerca di svolgere il proprio ruolo e di onorare la carica e l'istituzione che rappresenta. Ma sapevamo che era un mero esercizio di stile, perché comunque non ci sarebbe stato neanche il tempo per parlarne, neanche per presentarli in Commissione, figurarsi in Aula. Questo mortifica il ruolo del Parlamento, mortifica il ruolo di questa Camera, che diventa un organo che ratifica, e non è questa la nostra funzione. in premessa, sulla metodologia con la quale stiamo lavorando da un anno a questa parte, non solo non possiamo che esprimere il nostro dispiacere, ma anche stigmatizzare questa prassi che non ci piace, non ci appartiene e non è corretta per la storia parlamentare della nostra Repubblica. questo provvedimento si espone a una serie di osservazioni, riflessioni e anche critiche molto pesanti. Alcune riguardano lo strumento attraverso il quale il Governo pensa di gestire l'immigrazione, rifuggendo sempre da quella che sarebbe la soluzione più semplice, e cioè avviare un percorso legislativo tradizionale; avviare un percorso legislativo tradizionale; mettere mano a una riforma, a un testo unico sull'immigrazione e, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, finalmente

in conseguenza di un evento di cronaca di particolare scalpore: abbiamo una legislazione che non è soltanto d'urgenza, ma è anche di sensazione, poiché si muove sull'onda di una sensazione, di un evento che stimola la produzione di un decreto-legge. Invece di fare quello che si dovrebbe fare, continuiamo ad assistere a normative introdotte tramite decreto-legge che scalfiscono in ordine sparso i diritti dei cittadini e delle persone, in questo caso degli immigrati; ancor peggio, in questo caso si va a incidere anche sui diritti dei minori non accompagnati che arrivano in Italia dopo viaggi della speranza, mettendo a rischio la propria vita, dopo essere stati trattenuti in centri di detenzione in condizioni inumane. Per tutta risposta, invece di trovare un'accoglienza che tenga anche conto della loro età giovanissima, vengono trattenuti nei centri in un regime di sospensione di diritti civili: chi è trattenuto in questi centri non è detenuto, ma non è neanche libero; si trova in una sorta di sospensione dei diritti civili che è francamente inaccettabile, con un tempo che va via via aumentando. In questo periodo di tempo il Governo, invece di cercare di capire cosa si può fare, come gestire, in che modo accertare l'età dei minori che arrivano in Italia senza accompagnamento, introduce un nuovo strumento che è affidato alla pura valutazione arbitraria, in senso letterale, dell'autorità di pubblica sicurezza. Non c'è quindi un parametro certo, ma si dice soltanto che l'autorità di pubblica sicurezza, quindi il questore,

può disporre che, ai fini dell'accertamento dell'età del minore non accompagnato, vengano eseguiti degli esami antropometrici con delle misurazioni, ivi compresi anche gli esami radiografici. Come lo dispone l'autorità che è amministrativa? Lo dispone e lo comunica alla procura, la quale dà la propria autorizzazione con un provvedimento specifico o addirittura in forma orale. Quindi siamo arrivati a dire e a pensare che si possa prevedere che il questore lo chieda e il procuratore della Repubblica lo autorizzi al telefono. Questo è uno svilimento dei ruoli e delle funzioni tanto del questore, quanto della procura. Ove ciò non bastasse, voglio anche ricordare che i trattamenti sanitari in Italia - siamo in Italia e queste leggi si applicano a tutti si applicano a tutti - possono essere disposti obbligatoriamente soltanto nei casi previsti dalla legge e mai quando essi possono nuocere alla salute del soggetto nei cui confronti vengono disposti. allora, qual è lo scopo di sottoporre a un trattamento sanitario come l'esame radiografico un minore che arriva non accompagnato in Italia e dichiara di avere una certa età. Lo Stato italiano, che ha previsto addirittura di estendere il tempo del suo trattenimento giorni, in questo lasso di tempo non è in grado di avviare un procedimento, di chiedere i documenti, di fare anche quelle verifiche che prevede la legge Zampa per stabilire

C'è anche un'altra questione che forse è passata un po' in sordina, ma che è ancora più grave, che è quella della lesione dell'esercizio del diritto per i soggetti richiedenti protezione internazionale. Tra le maglie della discussione alla Camera, sono state inserite delle norme che hanno ulteriormente aggravato il testo e hanno limitato l'esercizio del diritto di difesa.

nuovi - il ricorso viene dichiarato inammissibile. Si ha così un'ulteriore conseguenza, ovvero che il soggetto nei cui confronti il ricorso viene dichiarato inammissibile perde anche il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio e il suo difensore, cioè quell'avvocato che si è onorato di presentare il ricorso, perde il beneficio alla liquidazione del compenso: cioè è come se lo Stato gli dicesse che la responsabilità è sua, ha proposto il ricorso ma non c'erano elementi nuovi e, quindi, ha lavorato e non ha diritto di essere pagato, neanche con il gratuito patrocinio. Questa è una lesione del diritto di difesa,. È una lesione di diritti civili. È una lesione macroscopica. È un sovvertimento dell'ordinamento giudiziario. È come dire che tutto diventa un arbitrio. Lo facciamo questo ricorso? E poi se ce lo bocciano? Bene, a quel punto perdiamo anche il diritto al compenso, come se il lavoro non fosse lavoro, come se la professione non fosse sempre meritevole di essere rispettata, anche quella dell'avvocato che difende i diritti civili dell'immigrato che chiede di essere ammesso alla protezione internazionale.

nella forma in cui lo stesso si esercita all'interno di uno Stato, decide di colpire una collettività, che siano dei cittadini, che siano dei portatori di interesse, che sia una eterogenea composizione di persone, agisce in due modi. Il primo nodo è attuare una legislazione specifica attraverso la quale vengono punite le condotte che quelle persone, la collettività che si vuole arginare e mortificare

decreto-legge si introduce la sanzione sostitutiva dell'espulsione per il minore che sia riconosciuto colpevole del reato di falsa dichiarazione di età. Questa è la norma speciale sulla norma speciale. Più discriminatorio di questo, signor Presidente, non c'è niente. Un cittadino italiano che fornisca infatti false generalità compie un reato e viene sottoposto alla pena prevista dalla legge; un cittadino straniero, immigrato irregolare, che fornisca una falsa dichiarazione sulla propria età e viene riconosciuto colpevole di questo reato, invece di scontare la pena prevista dal codice penale,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire con grande forza che oggi siamo chiamati di nuovo a votare l'ennesima questione di fiducia

vorrei discuterne con voi non perché ho le ragioni in tasca, ma perché siamo al quarto decreto-legge sull'immigrazione e non abbiamo risolto niente. Nulla è stato risolto. Possiamo discutere insieme? Il primo decreto affrontava la questione delle ONG: si volevano

questo terreno. Siete andati a Cutro e avete definito un decreto-legge Cutro, in spregio a una catastrofe avvenuta, a un naufragio. Ebbene, che cosa avete fatto? Avete abolito la protezione speciale.

provocano il degrado e addirittura la delinquenza e via dicendo. A

A voi sembra normale che, ad esempio, molte aziende funzionino grazie all'immigrazione? Tuttavia, se c'è l'immigrazione, è possibile fare un ragionamento in cui si discute di di condizioni sociali? Ad esempio, le imprese devono solo utilizzare la forza lavoro come manodopera o si devono preoccupare anche di dare un tetto a quei lavoratori e quelle lavoratrici? Si devono preoccupare e ci dobbiamo preoccupare di sviluppare la formazione, l'insegnamento, la scuola? Altrimenti, è certo che, oggettivamente, se si vive nel degrado,

Questo è il dato fondamentale. Per questa ragione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo estremamente convinti e abbiamo presentato anche una mozione di incostituzionalità, perché pensiamo che queste misure siano anticostituzionali.

non abbiamo risolto nessun problema; addirittura adesso pensiamo di decentrare i centri di detenzione - come li chiamo io - in Albania,

sicuritario, cioè sostanzialmente di controllo. Mentre invece - insisto - la necessità è come si fa l'inclusione; come si fa in modo che chi produce e contribuisce a produrre ricchezza si senta e diventi cittadino italiano;

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, comprendo che vi siano idee diverse e quindi anche sensibilità e polemiche su questo tema, che è uno dei temi più delicati e controversi del dibattito politico, culturale e sociale internazionale: il tema dell'immigrazione. Dico, però, ai colleghi che, alla fine, non possono immaginare che le elezioni e un Governo di un certo tipo non abbiano comportato un diverso orientamento sulle materie dell'immigrazione, dell'integrazione e delle sue modalità delle politiche di sicurezza. Questo provvedimento non dovrò nemmeno descriverlo nei dettagli, perché è stato al centro di tante discussioni. Purtroppo noi siamo in seconda lettura e - come accade a volte ai colleghi della Camera - le approfondite discussioni in prima lettura sacrificano la Camera che arriva dopo. Succede anche alla Camera sui provvedimenti che affronta il Senato. C'è un problema complessivo di funzionamento dei lavori parlamentari, sul quale è lecito riflettere; da qui le fiducie, da qui tutte le cose che oggi sono state dette che hanno anche un fondamento rispetto alla dinamica e alla vita parlamentare. Tuttavia, è un dato di fatto che il fattore politico della diversità delle impostazioni c'è, e noi non lo nascondiamo dietro un dito. Noi abbiamo su questa materia una lunga storia, perché il fenomeno si è accentuato e la movimentazione dei popoli nel pianeta si è accelerata negli ultimi trent'anni. La legge Martelli, che per molto tempo ha regolato questa materia, risale agli anni Novanta. Ricordo poi la legge Turco-Napolitano, con Giorgio Napolitano ministro dell'interno e Livia Turco ministro

con qualche articolo. Mi direbbero: «Eh, che orrore!». Ma anche la legge Turco-Napolitano conteneva molte vicende discutibili, dal nostro punto di vista, e altre che potrebbero oggi essere considerate perfino troppo severe. Poi c'è stata la legge Bossi-Fini, che per molti versi è ancora in vigore e che era una legge più severa. Però vorrei ricordare - questa cosa si è ripetuta anche adesso che a volte la sinistra fa le polemiche, dicendo che abbiamo fatto le grandi sanatorie. Quando si fece la legge Bossi-Fini, fu consentita la regolarizzazione di un numero enorme di stranieri presenti in Italia. C'era il problema delle badanti, più grave di quanto sia oggi, quando ormai ha assunto una sua dimensione fisiologica; allora era quasi una novità che ci fossero persone, provenienti da vari Paesi, che assistevano le persone anziane. Addirittura ci furono delle norme per evitare i matrimoni di comodo. Bisogna ricordarsi la legislazione, perché a volte, nei confronti dell'anziano italiano, c'era il tentativo facile che l'assistenza portava a un'affettività e poi casomai il matrimonio era strumentale per ottenere il permesso di rimanere in Italia, magari si acquisivano anche i diritti patrimoniali ed ereditari. Sono tutti dibattiti che ci sono stati in questo Paese, cari colleghi, e quindi non stiamo arrivando da Marte.

A volte le ragioni di schieramento non consentono quello che dovrebbe essere normale in un Paese: se si condivide un provvedimento altrui, lo si fa con la libertà del proprio mandato parlamentare. È però andata come è andata. Oggi c'è una politica molto equilibrata. Ho citato prima quella regolarizzazione che avvenne ai tempi della legge Bossi Fini. Il Governo in carica ha fatto un piano triennale che supera le 400.000 unità e non vi nascondo che, di fronte a quel numero, io stesso ho avuto qualche perplessità. perplessità. È vero che le associazioni di categoria e quelle agricole dicono che serve la manodopera; ma non vorrei che poi, in alcuni casi, la manodopera che arriva serva per calmierare il costo del lavoro, grazie a fenomeni di sfruttamento, che vanno combattuti, e di lavoro nero, oppure attraverso l'accettazione di condizioni salariali diverse. Se uno viene da zone poverissime, in condizioni di fame, è ovvio che già il fatto di arrivare in Italia a lavorare lo porta ad accettare condizioni salariali diverse da quelle di un nostro nostro connazionale, che sta qui dalla nascita, da sempre, e richiede una serie di riconoscimenti diversi. Occorre quindi fare attenzione, perché a volte ampliare troppo gli ingressi può favorire fenomeni di sfruttamento. Non voglio fare la polemica su quelli che poi si sono autorganizzati. Non so se i parenti dell'onorevole Soumahoro sono innocenti o colpevoli: non emetto sentenze. Abbiamo però visto che anche gli stranieri si organizzano: la cooperativa, l'associazione, è tutto in regola, quella casa va bene, l'assistenza è adeguata. C'è quasi una forma di autorganizzazione e dei fenomeni discutibili: definiamoli discutibili, poi saranno accertati, dove saranno accertati. Quindi, questo è il problema e il Governo ha dato spazio, con una programmazione triennale, ad oltre 400.000 ingressi: non ricordo nemmeno il numero esatto, ma è superiore. Dopodiché, il provvedimento in esame si inquadra in una politica complessiva. Il Piano Mattei riuscirà o non riuscirà? Risolvere i problemi dell'Africa e della sua esplosione demografica non è compito di un solo Stato. L'Italia ha il dovere di affrontarli, perché è nel Mediterraneo e ha una sensibilità. È stato questo Governo, con il presidente del consiglio Meloni e il ministro degli affari esteri Tajani, che ha convocato alla Farnesina i Paesi africani, per una politica di solidarietà, di aiuto e dialogo *(Applausi)*, e non per una politica di repressione o di razzismo. Dopodiché, ci vuole l'Europa, ci vuole il mondo e i soldi vanno spesi bene: non è che il problema dell'Africa lo risolviamo solo noi italiani, che abbiamo già tutti i problemi dei contratti, dei medici, della pensione e dell'occupazione. Ne abbiamo

Stiamo facendo un piano di aiuti alla Tunisia e alcuni esponenti dell'Unione europea di sinistra hanno rallentato quelle erogazioni. Di questo do anche una lettura politica: si discute tutte le volte sugli alleati del centrodestra, ma io discuto del boicottaggio di alcuni socialisti dell'Unione europea delle politiche di aiuto alla Tunisia *(Applausi)*. Ciò è più scandaloso di Tizio o Caio che, per carità, sono distinti e distanti da noi del Partito popolare europeo, ma credo che Fratelli d'Italia e la Lega siano partiti che governano l'Italia e sono pronti a fare la loro parte, in un quadro alternativo alla sinistra, in Europa. Quindi, onorevoli colleghi, stiamo facendo una politica di aiuto, di apertura, di dialogo e anche di maggiore fermezza. A proposito anche del controllo maggiore sui minori: quanti vengono fatti entrare passandosi per minori? Tutti a piangere dicendo che non si fanno sbarcare minori; poi, però, quando quei minori, se donne o uomini, vengono mandati sulle strade, a prostituirsi o a fare reati, nessuno si commuove più. *(Applausi)*. Essere più attenti vuol dire anche prevenire fenomeni di sfruttamento di tanti minori che finiscono in condizioni

come obiettivo. Invece fate entrare tutti, ma poi ci si gira dall'altra parte se in una campagna della Capitanata o in una fattoria della Sicilia o in una periferia di Roma o Milano un lavoro agricolo viene fatto da un lavoratore sfruttato o una donna viene fatta prostituire o se ad un bambino vengono fatti vengono fatti commettere crimini, perché poi ci sarà l'impunità, in quanto minorenne. Dovete preoccuparvi anche dopo della fine che fanno le persone che entrano. votiamo convintamente a favore di questo decreto-legge: misure più severe sul controllo dell'età dei minori, maggiori poteri alle autorità di polizia, i temi della sicurezza e le procedure di espulsione, che sono complicate - lo sappiamo bene - perché non sono questioni che si risolvono facilmente. Io non ho una visione "teologica" della legge, altrimenti basterebbero i dieci comandamenti e tutto funzionerebbe bene. Le leggi si fanno nella speranza che migliorino le situazioni. Alcune hanno funzionato, altre non hanno funzionato. Vado alla conclusione. Noi facciamo una politica di grande accoglienza, ma anche di maggiore severità. Abbiniamo piani per l'Africa al controllo delle nostre frontiere. Vogliamo essere solidali e non fare sfruttare quelle persone in maniera cinica, ma ne vogliamo fare entrare un numero programmato. Vogliamo dialogare con la Tunisia, con la Libia, con l'Egitto e con chiunque, perché il mondo è quello che è, e non è quello che noi sogniamo. Quindi, votiamo con convinzione questo decreto-legge e la fiducia al Governo, augurandoci - colleghi, dovreste farlo anche voi che queste norme funzionino. Ne ho elencate tante, il bilancio si farà in sede storica. Queste sono norme che noi condividiamo e che speriamo possano abbinare la solidarietà possibile con la sicurezza necessaria. Per questo - ripeto - votiamo a favore di questo decreto e la fiducia al Governo.

contrariamente a quanto è stato poc'anzi detto, questo decreto-legge è lo specchio della totale incapacità e disperazione del Governo rispetto al fenomeno della migrazione.

disperazione perché sono di fronte alla loro incapacità di tenere fede alla propaganda fatta durante la campagna elettorale. *(Applausi)*. Oggi assistiamo, come fa un pipistrello che sbatte contro le pareti di una stanza chiusa, alla ricerca alla ricerca di una via d'uscita. Ma la loro incapacità è stata certificata dalle stesse parole della *premier* Meloni, la quale, per sua stessa ammissione, ha detto che che in Europa non le rispondono neanche al telefono. Da qui il totale fallimento delle politiche che cercano di mettere in atto. Un'altra delle conseguenze a cui abbiamo assistito in questi giorni è stata l'umiliazione che Roma, la mia città,

quando anche quella votazione dimostra invece l'assoluta inconsistenza del peso politico dell'Italia di Meloni sulla scena internazionale. Veniamo a questo decreto, che calpesta tutto ciò che si può calpestare, tutto ciò, anzi, che non si dovrebbe mai calpestare: la Costituzione, i Regolamenti di Camera e Senato, i diritti umani, le convenzioni internazionali e, in ultima analisi, la ragione stessa. Mai come in questo decreto-legge le questioni di metodo e di merito sono inestricabilmente intrecciate. Il metodo Il metodo è portato avanti con la violazione della Costituzione: noi siamo anche stanchi di ripetere la violazione dell'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, perché voi siete andati oltre il monocameralismo, voi siete arrivati al mezzo cameratismo. Voi, infatti, avete umiliato anche la Camera, contingentando i tempi di esame di questo decreto alla Camera. Al Senato è arrivato ieri in Commissione. Oggi vola qui in Aula con il voto di fiducia: tempi di approfondimento, zero. Infatti, i risultati si vedono. *(Applausi)*. Su questo torneremo, ma dicevo che il metodo si intreccia quanto mai con il merito, perché qui il metodo ha delle ricadute dirette sulla violazione dei diritti umani e in particolare sulla violazione dei diritti umani dei minori, che voi, con questo decreto, istituzionalizzate. Faccio notare che è con questo stesso atteggiamento autoritario che questa maggioranza e questa compagine governativa vorrebbe mettere mano, vorrebbe manomettere, la Costituzione repubblicana. È di ieri pomeriggio la notizia della condanna dell'Italia da parte della da parte della Corte europea dei diritti umani rispetto al trattamento dei minori. «Italia bocciata sui minori»: così apre il giornale «Avvenire».

nell'*hotspot* di Taranto. Quando? Nel 2017. Ora, si parla di analfabetismo funzionale quando da un testo non si riesce ad estrapolare l'informazione principale, distinguendola dalle informazioni accessorie. L'informazione accessoria è al 2017. L'informazione principale è che non si possono detenere i minori insieme agli adulti nei CPR e voi, con questo decreto, ce li detenete non per due mesi, come nel caso di Taranto, ma per cinque mesi e lo mettete per iscritto!

di più. Ho dovuto sentire parole secondo le quali tutto questo viene fatto a tutela dei minori. Allora, a tutela dei minori, da oggi, in base alle volontà di questo Governo, l'Italia misurerà, anche attraverso radiografie, attraverso esami antropometrici, le ossa, la circonferenza toracica. L'Italia farà esami sanitari: ai

i maggiorenni che arrivano in Italia e si dichiarano minorenni. Innanzitutto, questo è falso. È falso, signor Sottosegretario, e lei lo sa. Rispondo anche al senatore Gasparri, che ha fatto una tirata retorica sostenendo che poi i minorenni finiscono nei campi, sfruttati dal caporalato, e le minorenni finiscono, purtroppo, come ben sappiamo, nel giro della prostituzione. È esattamente il contrario. Il pericolo è che i minorenni che arrivano in Italia, come succede la maggior parte delle volte, si dichiarino maggiorenni appositamente per poter lavorare perché vengono qui per lavorare ed è così che finiscono nelle reti dello sfruttamento, sessuale e lavorativo. Quindi, è esattamente il contrario di quello che fate voi. La previsione contenuta in questo decreto, di misurare le persone antropometricamente, addirittura utilizzando utilizzando i raggi X, davvero ricorda altri tempi. Ricorda altre misurazioni, in cui l'essere umano veniva catalogato in base, appunto,

le misurazioni degli animali. È inutile che si dica che sono strumenti che in parte sono già in vigore. Allora andrebbero aboliti, perché sono strumenti inumani e degradanti; andrebbero aboliti, mentre li sostenete, li ampliate *(Applausi)* e li volete usare sui minori: questa è la cosa che più desta sconcerto.

veramente una follia, una cosa assolutamente senza senso, come l'intero decreto-legge, che - lo ripeto - è frutto della disperazione e della vostra incapacità di gestire un fenomeno purtroppo strutturale, perché il dato di fatto che rimane è che voi

il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, non può votare la fiducia ad un Governo che calpesta la Costituzione, il Parlamento, i diritti umani e i minori. iscritto a parlare il senatore Guidi.

che rappresenta per noi un'emergenza soprattutto in questo periodo, in cui ci sono fattori esterni che hanno accelerato l'arrivo nel nostro Paese di immigrati irregolari. quindi convinti che la decretazione d'urgenza sia uno strumento opportuno per affrontare quella che per noi - lo ripeto - è un'emergenza, a differenza di qualche altra forza politica che ritiene che questo fenomeno rappresenti un'opportunità. Quindi sì alla decretazione d'urgenza, che non ci scandalizza; anzi riteniamo che bene abbia fatto il Governo nel corso di questo anno di legislatura a intervenire per ben due volte e, se sarà necessario, anche nei prossimi anni, perché è un fenomeno in evoluzione che necessita di continui aggiornamenti delle normative, di correzioni, di adeguamento alle fasi in cui questo fenomeno va modificandosi. Quindi fa bene il Governo a intervenire con correttivi puntuali laddove, per l'esperienza sul campo degli uomini dello Stato, si renda necessario farlo costantemente. Per quanto ci riguarda, si tratta di interventi importanti, ma evidentemente non sufficienti; sappiamo anche noi che non sono sufficienti, perché è un fenomeno di tale portata che

in fase di crescita costante e molto preoccupante; un fronte nuovo rispetto ai flussi provenienti da altre parti del Mediterraneo, dalla Libia in particolare. I dati danno ragione al Governo: ci sono dei cali grazie all'accordo voluto dal Governo italiano con la Tunisia. Da soli, come sempre, abbiamo affrontato questo tema e lo stiamo affrontando in modo efficace e nessuno può controvertere questi dati, che sono un fatto reale reale e acquisito. Il tema dell'immigrazione, a differenza della sinistra, per noi va gestito, governato, per cui servono regole non solo in Italia ma anche a livello europeo. Rigettiamo al mittente tutte le accuse che sono state mosse dalla sinistra quest'oggi e in passato, che a nostro avviso evidenziano solo la differenza che esiste tra la nostra impostazione, quella del centrodestra e della Lega, nell'affrontare questo tema e l'impostazione delle forze della sinistra. È stato detto che questo decreto-legge aumenta la clandestinità. Ma io chiedo: qual è la risposta della sinistra? Se portassi agli estremi le vostre posizioni, potrei ritenere legittimamente, dalle parole che voi pronunciate in ogni occasione, che a vostro avviso chiunque arrivi in Italia debba ricevere la legittimità a soggiornare nel nostro Paese senza limite di sorta. Noi riteniamo, invece, che debbano esistere debbano esistere delle regole e che vadano applicate, che le forme di espulsione vadano rafforzate, che i rimpatri vadano perfezionati e quindi diciamo sì anche per questo motivo a questo decreto. Si dice anche, da parte della sinistra, che serve manodopera, che servono lavoratori. Lo diciamo anche noi, ma con flussi regolari e la dimostrazione che questo Governo è coerente è quel provvedimento che è stato citato anche dal collega Gasparri, che prevede un aumento di quote di flussi regolari per dare una risposta di manodopera alle nostre imprese, a chi lavora nel turismo, ma nell'agricoltura e che avanza queste richieste. Noi crediamo nella regolarità dei flussi, non nell'afflusso irregolare nel nostro Paese, che spesso e volentieri non è indirizzato al lavoro, ma anche ad altre attività fatte di espedienti sul nostro territorio. Questo decreto stabilisce un criterio chiaro: chi delinque non è gradito nel nostro Paese e va espulso. Diciamo quindi sì anche per questa ragione agli articoli che sono stati presentati dal Governo in questo decreto.

anni. È evidente che è un numero enorme, che spinge a ritenere legittimamente che alcuni di questi minori effettivamente non lo siano, che si

migranti maggiorenni, un costo per le nostre comunità, per i Comuni e per lo Stato e quindi è giusto e corretto che il Governo intervenga in questo decreto per stabilire chi veramente è minore e chi non lo è. Questo, fra l'altro, perché l'accertamento dell'età non è certamente un intervento invasivo e già esiste, è stato già chiarito anche questo aspetto. C'è un altro elemento che ci distingue dalla sinistra. Noi riteniamo che purtroppo flussi irregolari di migrazione aumentino la criminalità nelle nostre città, nelle nostre comunità. Lo dicono i dati

noi e ai cittadini, è solo la sinistra che continua a parlare di una distorta percezione della sicurezza, come se come se questi episodi che accadono ormai quotidianamente nelle nostre grandi città in particolare vadano ormai accettati come impossibili da evitare, come una condizione a cui ci dobbiamo adattare. Ebbene, noi non ci adattiamo alla criminalità dilagante all'interno delle nostre città e alle situazioni di degrado, quindi riteniamo necessario e opportuno che il Governo intervenga e in questo decreto ci sono alcune risposte: le nuove unità di militari dedicati al progetto «Strade sicure» che il Governo PD e Cinque 5 Stelle aveva depotenziato in modo irreparabile; altri interventi che finanziano gli straordinari per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; l'acquisto di beni strumentali per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Si tratta di risposte concrete all'emergenza sicurezza e gestione dell'immigrazione. I numeri dell'immigrazione ci preoccupano perché il nostro Paese non è in grado di gestire questi numeri, non lo è il Governo, ma non lo sono nemmeno le comunità e gli enti locali di qualunque colore politico, che chiedono al Governo di farsene carico. quindi giusto che il Governo intervenga a livello nazionale, con una legislazione costante e coerente con il fenomeno, che va aumentando, e agisca a livello internazionale. Questo Governo sta facendo una cosa e l'altra con il massimo dell'impegno. Chi è assente in questa partita, a parte la sinistra - ripeto - per la quale il fenomeno non va gestito, non va controllato, ma semplicemente accettato? È l'Europa, che forse solo negli ultimi tempi - quantomeno a parole - ha deciso di intervenire. Vi è poi un problema di fondo: l'immigrazione è un'opportunità o rappresenta anche un problema per il nostro Paese? Con i numeri attuali è un problema. Per la sinistra non lo è, tanto è vero che ho sentito dire anche oggi che l'immigrazione è la risposta al calo demografico degli italiani. Noi non accettiamo questo teorema, non accettiamo l'idea che l'Italia debba diventare un Paese popolato a maggioranza da immigrati. L'accoglienza e l'integrazione sono giuste, ma è necessario che l'Italia - e noi crediamo in questo - rimanga il Paese degli italiani, non degli immigrati. Diciamo no alla distruzione della nostra società e del nostro modello culturale, che per noi rimane un valore da coltivare e difendere. La sinistra italiana ed europea non la pensa allo stesso modo,

Signor Presidente, «tre volte indifesi perché minori, perché stranieri, perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra di origine e separati dagli affetti familiari».

Tre volte indifesi perché minori, perché stranieri, perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra di origine e separati dagli affetti familiari. Tornerò su queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel gennaio 2017, qualche mese prima che la legge n. 47 (che io preferisco chiamare così; sono orgogliosa di aver

Una legge che oggi voi di fatto smantellate per coprire il fallimento delle vostre politiche in materia di immigrazione.

non solo per lo schiaffo - l'ennesimo - che il Governo Meloni assesta al Parlamento e alla sua stessa maggioranza; dovreste essere voi i primi a indignarvi per come sta funzionando la democrazia e per come venite trattati. Ieri, in Commissione, vi abbiamo ascoltato infatti ammettere di fronte a noi che non avete avuto nemmeno il tempo di leggere queste norme. *(Applausi)*. E si capisce da quello che dite in quest'Aula che non le avete nemmeno potute leggere. Non Non solo per noi che crediamo nella capacità di questo Paese di costruire una risposta all'altezza della sfida più complessa del futuro, quella della migrazione; fenomeno strutturale che non ha più nulla di emergenziale.

nulla di rispettoso del diritto su cui è stato edificato lo Stato italiano. Questo, però, è un giorno profondamente triste per chi difende i diritti umani, a partire da quelli che tutelano le persone di minore età indicate nella Convenzione di New York, sottoscritta e ratificata dall'Italia; è un giorno triste per i destini di quei ragazzi che attraversano a piedi Paesi interi, con mezzi di fortuna, mettendo a rischio la propria vita, subendo violenze indescrivibili,

convinte di venire a lavorare in Italia o in un altro Paese europeo che loro sognano accogliente e si trovano, invece, a subire ogni genere di sfruttamento, a partire da quello fisico e sessuale. Queste norme sono gravi, calpestano la Costituzione, colpiscono lo Stato di diritto laddove, ad esempio, si prevedono misure restrittive sul diritto di difesa del soggetto espulso, in violazione di ben tre sentenze della Corte costituzionale. in esame resterà nella storia per la sua inedita volontà politica di colpire i fragili e gli indifesi, di cui il Papa parlò al mondo e alle istituzioni politiche, sperando - io credo che lui lo sperasse di far comprendere a tutti che le migrazioni oggi non sono un fenomeno limitato ad alcune aree del pianeta, ma toccano tutti i continenti e vanno sempre più assumendo le dimensioni di una drammatica questione mondiale e che sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell'emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla miseria, dalle condizioni ambientali, fattori a cui si associa anche la globalizzazione nei suoi aspetti negativi. Ogni studio, ogni analisi pubblicata da organizzazioni internazionali di tutela dell'infanzia per l'infanzia e l'adolescenza, al termine di una lunga indagine conoscitiva, hanno certificato che quelle ragazze e quei ragazzi arrivano alla ricerca di una vita migliore per sé, ma intenzionati anche ad aiutare la madre o i fratelli rimasti a casa, ignari dei pericoli enormi che li attendono nei viaggi infiniti e pieni di un coraggio che colpisce. Non tutti ce la fanno. Io porto con me da anni la foto di due bambine, una siriana e una palestinese, tanto simili fisicamente che il nonno della piccola partita dalla Siria con la famiglia, non avendo mai più avuto notizia di nessuno di loro, informato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) del lavoro che andavamo facendo sui minori migranti, si mise in contatto con me, sperando che fossero la stessa persona, dato che una risultava sbarcata da sola in Sicilia. Purtroppo non era così: la piccola siriana era morta in mare con i fratelli. Per la palestinese io conto, so che ha trovato e abbia potuto trovare una famiglia accogliente, un tutore volontario, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, che al momento della sua approvazione suscitò una risposta straordinaria nella società italiana: in poco tempo e con minima pubblicità si iscrissero all'albo dei tutori e delle tutrici volontari oltre 5.000 persone, per lo più donne. Li abbiamo ascoltati, li abbiamo incontrati, li abbiamo visti arrivare ai confini del nostro Paese e ai confini dell'Europa. Ad oggi il numero complessivo di bambini, bambine e adolescenti non accompagnati presenti in Italia risulta di circa 23.000, con una forte presenza di minori che provengono dall'Egitto, dall'Ucraina, dalla Tunisia, dalla Guinea, dal Gambia, dalla Costa d'Avorio e dall'Albania. Quello stesso Paese a cui chiedete di aprire centri di detenzione per i migranti che arrivano da noi, in una sorta di subappalto delle vite umane, una cosa grottesca: 23.000-24.000 minori, in un Paese che rientra tra le dieci potenze del mondo, di fronte ai quali gettate la spugna e certificate il fallimento delle vostre stesse politiche. Erano 25.000 nel 2016, quando, spinto dalla volontà di dare una risposta che facesse onore al Paese e alla sua storia (lo dico a voi, che vi presentate come patrioti) e che ci facesse stare con onore nei consessi internazionali a discutere di diritti dei migranti e dei minori migranti, il Parlamento italiano, con una larghissima convergenza tra le forze politiche tutte, approvò quella legge, scommettendo sulla capacità di accogliere questi giovani, come un'opportunità in un Paese che invecchia, che è già invecchiato, che stenta a trovare le risorse necessarie per il sistema produttivo, per sostenere il sistema pensionistico, per costruire una società capace di convivere. Il sottosegretario Molteni ha detto che era necessario un tagliando e lo ha ribadito più volte; ho tremato la prima volta che gliel'ho sentito dire. Convengo con lui, però: era necessario un tagliando. Tuttavia era necessario per implementare la realizzazione delle misure previste dalla legge, non per demolirla. E allora mi domando, se era necessario questo, perché avete smantellato lo SPRAR? Perché avete smantellato un sistema di accoglienza diffuso che funzionava? Perché non avete cominciato voi a realizzare i CAS dedicati? Perché non avete aumentato i posti nel SAI e nel FAMI? No, lo si poteva fare, perché è molto più facile cambiare le norme sul riconoscimento dell'età, mettere questi giovani per un tempo lunghissimo in un limbo senza senso, quello dei centri, in promiscuità con gli adulti, dove voi non mettereste mai un vostro figlio o un vostro nipote. Mai. Tanto che cosa importa? Sono stranieri. Questo oggi si è capito dai vostri interventi in quest'Aula: esistono due specie di esseri umani, gli stranieri e quelli che non sono stranieri. Solo questo avete dimostrato oggi. State approvando norme che disonorano questo Paese e certificate il fallimento della vostra politica. Torno a dare la parola a Papa Francesco e concludo: ognuno è prezioso, le persone sono più importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul modo in cui tratta la vita e la dignità dell'essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori migranti. Bene, noi su questo vi misuriamo ed è per questo che votiamo "no" convintamente a questo decreto. Signor Presidente, membri del Governo, cari colleghi umani e non umani (perché ormai siamo distinti tra categorie di umani e non umani) umani) e futuri candidati alla Corte costituzionale (visto che sono diventati tutti i costituzionalisti e sanno tutti per certo che qualsiasi norma facciamo in qualsiasi momento è incostituzionale), questo decreto-legge interviene su alcuni temi che ovviamente sono stati completamente ignorati dalle opposizioni, perché fa loro comodo ignorarli. La misura delle offese che sono state pronunciate in Aula la dice lunga sulla volontà di approfondire veramente questo decreto. Tutta questa volontà di approfondirlo forse non c'era. E vi dico anche che non siamo stati noi in Commissione a dire di non aver letto il decreto, ma è stato qualcun altro dell'opposizione. Noi il decreto lo abbiamo letto, nonostante il poco tempo; voi evidentemente no, altrimenti ci avreste spiegato il motivo per il quale siete contrari al fatto che impediamo che entrino sul nostro territorio a persone che mutilano altre persone *(Applausi)*, persone che gettano l'acido in faccia e distruggono la vita di altre persone, persone che fanno lesioni superiori ai venti giorni a disabili e incapaci. Ci avreste spiegato il motivo per il quale siete contrari all'accelerazione delle espulsioni delle persone che sono pericolose per il nostro territorio *(Applausi)* e per la sicurezza del nostro Stato. Ci avreste spiegato perché siete contrari al fatto che questo Governo metta fine alle domande reiterate in continuazione per paralizzare l'azione delle istituzioni Siete contrari al fatto che ci siano delle persone che prendono in giro lo Stato italiano e si approfittano del fatto che lo Stato italiano accoglie tutti, ma non siamo disponibili ad accogliere i criminali, non siamo disponibili ad accogliere chi non ha titolo per entrare sul nostro territorio *(Applausi)*, non siamo disponibili ad accogliere le persone che sono un pericolo per la sicurezza. inumani, senza cuore, cattivoni, l'*evergreen* dei nazifascisti, perché quello è un *evergreen* che va sempre bene. Cari colleghi, ho già provato a dirlo non mi ricordo neanche quanto tempo fa: tempo fa: voi e nessun altro qua dentro può dare patenti di umanità agli altri. *(Applausi)*. Nessuno lo può fare e dovreste avere la decenza di stare in silenzio su questo, perché gli unici che hanno avuto una certificazione di inumanità siete voi, nel 2017, quando governavate. *(Applausi)*. Oggi fate le prediche sull'umanità, ma gli unici che hanno avuta la certificazione a Strasburgo siete voi e governavate anche nel 2016 e nel 2015, salvo che non vogliate dare la colpa al primo Governo Berlusconi per la vostra certificazione di inumanità. Magari qualcuno ci crede nelle vostre sedi del PD, ma non altrove. Allora vi dico che la verità è davvero molto semplice e gli italiani l'hanno capita bene: da una parte c'è chi vuole gestire il fenomeno dell'immigrazione, chi vuole mettere delle regole e frenare l'immigrazione clandestina che genera i morti in mare. Ripeto: più barconi partono, più morti in mare ci sono; purtroppo questa è la realtà statistica C'è chi vuole contrastare gli scafisti e vuole gestire il fenomeno che è in una fase emergenziale; dall'altra parte, mi dispiace dirlo, c'è una sinistra ipocrita e ignava, perché questa è la verità, che nel corso degli ultimi dieci anni è stata complice dell'immigrazione illegale, perché girarsi dall'altra parte di fronte a fenomeni di illegalità così diffusa è essere quantomeno ignavi. ignavi. Odiare il fatto che esistano dei confini ha danneggiato questo Paese; pensare che la parola "stranieri" sia una parolaccia (come ha detto, ha detto, in modo molto garbato, il senatore Delrio: non chiamiamoli stranieri) parte proprio dalla logica distorta del fatto che esistano dei confini. Voi li odiate i confini, noi invece i confini li vogliamo difendere. *(Applausi)*. legittimo pensare di difendere i confini, così come credo che sia legittimo pensare che, se si vuole veramente accogliere, bisogna farlo con qualità. Certo, l'emergenza diffusa ha funzionato e molte cooperative dicono che ha funzionato molto bene per i loro bilanci. Dobbiamo essere sinceri. io non ho capito però qual è la soluzione che viene proposta, perché ho sentito tante offese, ma poche soluzioni.

siete andati di fronte ai CPT e ai CPR, che voi avevate creato, con le bandierine della pace, dicendo che lì c'erano trattamenti inumani e avete iniziato a chiuderli sul territorio.

avete fatto una sanatoria costante sul nostro territorio. Era necessario, dunque, era indispensabile ripristinare le regole. Ed è il motivo per il quale siamo intervenuti sui permessi di soggiorno reiterati, vi prendevano e ci prendevano in giro come Stato, quelli che erano clandestini e che restano clandestini. Avete distrutto gli accordi internazionali. Avete provato anche a boicottare e distruggere quelli fatti dall'Italia. Un accordo internazionale buono esisteva, che non avete distrutto.

uno straordinario esempio di cooperazione, che questo Governo vuole riprendere e che ha ripreso, ad esempio, con l'Albania. Evidentemente è un modello che a qualcuno piace,

E vi dico che noi saremo analfabeti funzionali, ma voi siete incompetenti istituzionali. Chi lo ha detto è un incompetente istituzionale e l'ha dimostrato nel precedente mandato. *(Applausi)*. Ma qual è, dunque, la soluzione che proponete ai problemi che vi ho illustrato prima? Non ce n'è stata una. Come pensate e come avreste pensato di agire nei confronti di questi farabutti che mutilano i genitali o fanno cose simili? Come pensavate di intervenire per accertare l'età di un minore? Ma come pensate che si faccia? Come pensate che facciano oggi i tribunali per accertare l'età di un minore?

minore o non è minore? Facciamo produrre le foto con le candeline della torta di compleanno per capire se è minore? Come vogliamo fare? Spiegatelo! Date delle soluzioni alternative! Non le avete date! A meno che a voi non vada bene che entri chiunque!

La vostra soluzione è sempre stata non dare una soluzione. Questa, purtroppo è la verità. È vero, è una questione di postura, come qualche collega ha detto. devo essere sincero, la vostra postura a me sembra un po' più da decubito *(Applausi)*, sono indeciso se prona o semiprona rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Sicuramente la nostra postura è eretta,

qualcuno pensa che li facciamo perché non sappiamo come intervenire, rispondo che l'Italia ci guarda con favore, perché fare tanti decreti-legge vuol dire che c'è la volontà di intervenire e di mettere una pezza ai danni fatti in passato. E i risultati...

I dati di ottobre e di novembre, rispetto a quelli del 2022 e del 2021, sono in calo. Poi voi potete raccontare tutte le scemenze... Senatore Lisei, le ho già concesso due minuti in più rispetto ai colleghi. La prego di concludere e di utilizzare delle terminologie consone. Un'altra cosa che le chiedo, e la chiedo a tutti i colleghi, è di rivolgersi alla Presidenza. Chiedo scusa ai colleghi per l'eccesso di *verve*, anche se mi interrompono in continuazione. Starò loro antipatico, evidentemente. Comunque è davvero antipatico Comunque è davvero antipatico essere insultati per un'intera discussione come è accaduto e non dover replicare alle accuse di inumanità, anche perché poi bisognerebbe capire qual è il vostro modello di umanità.

dell'umanità. Ribadisco che, di fronte all'emergenza dell'immigrazione, abbiamo scelto di scegliere, abbiamo deciso di decidere e ci siamo determinati di determinare, di bloccare le migrazioni clandestine...

quindi di concludere. LISEI *(FdI)*. Abbiamo deciso di decidere e non saremo ignavi come chi ci ha preceduto. Ci hanno votato per fare questo e il mandato degli elettori non lo tradiremo. nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 951, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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 Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Manca.

Gasparri,

2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge